Grazie Grazie

del Governo, il Documento di economia e finanza che ci occupa è il primo dell'attuale Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma del prossimo triennio. Questo Documento conferma le principali direttrici dell'azione di Governo che, com'è noto, si basano sul rafforzamento della rete di protezione e inclusione sociale, sulla semplificazione e sull'efficientamento delle politiche fiscali, sulla riduzione progressiva del differenziale di crescita del nostro Paese rispetto a quello della media dell'Unione europea, nonché sulla riduzione del rapporto debito/PIL. Questi obiettivi saranno raggiunti mediante il rilancio degli investimenti, il sostegno alle imprese per l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica, l'aumento complessivo della produttività, la riforma fiscale che renda il fisco più equo, più sostenibile e più semplice e, infine, il rafforzamento delle politiche sociali e del lavoro. Il rallentamento dell'economia globale, rilevabile in circa il 70 per cento dei Paesi, come indicato dal Fondo monetario internazionale, è principalmente riconducibile all'acuirsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, alla perdurante incertezza legata alla Brexit, all'accresciuta instabilità socio-economica all'interno di alcune economie emergenti; tutto ciò ha fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e dei mercati finanziari e, di conseguenza, ha influito negativamente sulle condizioni di scenario economico internazionale in cui si colloca l'azione di Governo per la nostra economia. La congiuntura internazionale ha causato una diminuzione della domanda estera, sia per l'Italia sia, in misura ancora maggiore, per la Germania, avendo queste due economie una spiccata vocazione all'esportazione, essendo rispettivamente il primo e il secondo Paese manifatturiero in Europa. In particolare, la crescita prevista del PIL italiano nel 2019 è, complessivamente, dello 0,2 in diminuzione rispetto alle previsioni della legge di bilancio. Ma, come detto, tale diminuzione è inferiore a quanto rilevato, ad esempio, per la Germania, che è passata da una previsione di crescita del 2,1

Il dato che riguarda l'Italia prende oggi atto della repentina e drastica mutazione del quadro internazionale, mentre non può dirsi che ci sia stato eccessivo ottimismo da parte del Governo nei mesi scorsi. Basti pensare che la Commissione europea, a novembre (quindi qualche mese fa) stimava per il 2019 una crescita all'1,2 per cento, mentre, nello stesso periodo, gli istituti indipendenti italiani stimavano uno 0,8 Del resto, i primi segnali di rallentamento del ciclo economico nell'area euro si erano evidenziati già nel 2018, quando si era calcolata una diminuzione della crescita del PIL, che si era attestata all'1,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2017. Infatti, anche in Italia nel 2018 l'economia aveva perso slancio, registrando una crescita del PIL reale dello 0,9 per cento, in discesa rispetto all'1,6 per cento registrato invece nell'anno 2017. In ogni caso, l'attuale livello previsto di crescita italiano tiene conto dell'aumento della domanda interna originato soprattutto dalla maggiore possibilità di consumo di oltre 5 milioni di italiani, ossia quei nostri connazionali che percepiranno il reddito di cittadinanza. In altri termini, con quel provvedimento abbiamo messo soldi nelle tasche di chi nulla aveva e questo, oltre a essere un provvedimento che va nella direzione dell'equità sociale e della lotta alle diseguaglianze, ha e avrà una funzione anticiclica, in quanto aumenterà la domanda interna; il che compenserà, almeno in parte, la diminuzione della domanda estera. Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2019 riflette, dunque, l'effetto di trascinamento negativo derivante dal rallentamento della crescita dell'economia italiana registrato già nel secondo semestre del 2018, in un contesto economico internazionale ed europeo risultato molto più difficile di quanto fosse possibile prevedere in autunno.

per gli anni successivi il DEF prevede prudenzialmente che il tasso di crescita reale si innalzi allo 0,8 per cento negli anni 2020, 2021 e 2022. Nel corso del 2019 ci sarà un impatto positivo sulla crescita congiunturale dei consumi delle famiglie - lo dicevo poc'anzi - che deriverà essenzialmente dal reddito di cittadinanza, a partire già dal secondo trimestre di quest'anno, e che stimolerà i consumi delle famiglie meno abbienti che, come noto, hanno una propensione al consumo più elevata della media. Ciò da solo sarebbe in grado di determinare un effetto positivo sulla crescita del PIL reale cento sia nel 2019 sia nel 2020. È appena il caso di accennare - ma su questo tornerà la collega Rivolta, che parlerà subito dopo - che è auspicabile un cambio di marcia nelle politiche economiche a livello europeo che stimoli la domanda interna di tutti i Paesi dell'Unione. Una crescita ai consumi, agli investimenti e, in definitiva, all'occupazione, deriverà anche dalla *flat tax* che sarà già in vigore nel 2019 per i piccoli imprenditori e per i professionisti, e di questo effetto si è tenuto conto nel DEF. Per ciò che riguarda le misure relative al sistema previdenziale (la cosiddetta quota 100, ma anche altro) dovrebbero avere un effetto neutrale quest'anno, mentre si attende un effetto positivo sulla crescita di circa 0,1 punti percentuali nel 2020. Anche le maggiori Anche le maggiori risorse per gli investimenti pubblici, stanziate dalla legge di bilancio 2019, dovrebbero fornire un ulteriore stimolo alla domanda già a partire dal secondo trimestre dell'anno, con un contributo alla crescita del PIL reale superiore allo 0,1 Nel nuovo quadro tendenziale dei conti della pubblica amministrazione, gli investimenti aumenterebbero del 5,2 per cento. Nel quadro programmatico dell'economia, che quindi sconta

I dati sia tendenziali sia programmatici sono stati validati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale ha evidenziato che le previsioni del DEF e le dinamiche del PIL reale e nominale si collocano nell'intervallo di variazione delle stime di riferimento. Per ciò che riguarda il calcolo relativo all'occupazione, le politiche del lavoro e della formazione connesse al reddito di cittadinanza faranno sì che tanti inattivi saranno considerati in cerca di lavoro, contrariamente a quanto succede ora, e il tasso di disoccupazione è previsto in discesa nel 2021 e nel 2022, tornando quindi ai livelli del 2018.

come già anticipato dal collega Marco Pellegrini, questo è il primo Documento di economia e finanza di questa legislatura, che traccia le linee di politica economica e di bilancio e delle riforme previste nel prossimo triennio. Il rallentamento della congiuntura in atto, principalmente riconducibile alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, congiunte all'emersione di tensioni geopolitiche in altri rilevanti Paesi e alla cresciuta instabilità socio-economica all'interno di alcuni Paesi emergenti, ha fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari. Ciò ha influito negativamente sulle condizioni dello scenario economico internazionale, in cui si colloca l'azione di Governo per l'economia italiana. Gli effetti del rallentamento si sono riscontrati sulla domanda interna dei principali Paesi, attraverso un sensibile calo degli investimenti e una moderazione L'attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla produzione dei beni d'investimento, ha subìto una battuta d'arresto, facendo risultare particolarmente esposti le economie altamente specializzate nel settore industriale ed i connessi Paesi ed i connessi Paesi fornitori di semilavorati. In particolare, per quanto riguarda l'area dell'euro, i primi segnali di rallentamento del ciclo economico si sono registrati già dal 2018, allorché si è registrata una diminuzione della crescita del PIL, che si è fermata all'1,8 per cento, rispetto al 2,3 per cento del 2017, venuta meno la spinta propulsiva del commercio estero. Come accennato, poiché la moderazione ha riguardato principalmente il settore manifatturiero, a fronte di una dinamica più resiliente dei servizi, ne sono risultati maggiormente interessati Paesi quali la Germania e l'Italia, le cui economie, come noto, sono a trazione industriale. Non solo: il clima di fiducia degli operatori economici europei e le relative scelte d'investimento sono stati fortemente condizionati anche dall'incertezza che ha accompagnato gli sviluppi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ancora in corso di definizione. Per l'Italia il Documento evidenzia come l'economia già nel 2018 abbia perso slancio, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,9 per cento in discesa rispetto all'1,6 per cento registrato nel 2017. Il fatto che ha maggiormente influito sul quadro congiunturale dell'economia nazionale è il netto ridimensionamento del contributo positivo della domanda interna e, in particolare, della componente dei consumi privati. Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2019 riflette dunque l'effetto di trascinamento negativo derivante dal rallentamento della crescita dell'economia italiana registrato già nel secondo semestre del 2018, in un contesto economico internazionale ed europeo più difficile di quanto previsto nello scorso autunno. Ad ogni modo per l'Italia, nel quadro tendenziale contenuto nel Documento, la previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2019 è rivista al ribasso di 0,9 punti percentuali, ossia allo 0,1 per cento, rispetto all'uno per cento prospettato nello scenario dell'ultimo documento di aggiornamento del quadro macroeconomico di finanza pubblica, presentato nel dicembre scorso nella Nota tecnica illustrativa annessa al bilancio 2019. Per gli anni successivi il Documento prevede prudenzialmente che il tasso di crescita reale si innalzi gradualmente allo 0,6 per cento nel 2020 e allo 0,7 per cento nel 2021, fino ad attestarsi allo 0,9 per cento nel 2022, mantenendosi per tutto il periodo previsionale al di sotto del profilo profilo tracciato nello scorso dicembre. In tal senso, indubbie sono le attese di un impatto positivo sulla crescita congiunturale dei consumi delle famiglie che deriverà dal reddito di cittadinanza a partire dal secondo trimestre di quest'anno, che dovrebbe fornire uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti che hanno chiaramente una propensione al consumo più elevata della media, che da sola sarebbe in grado di determinare un effetto positivo sulla crescita del PIL reale di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 che nel 2020. In termini analoghi, si stima che le misure relative al sistema previdenziale (la cosiddetta quota 100) dovrebbero avere un effetto neutrale quest'anno, mentre si attende un effetto positivo sulla crescita del livello del prodotto di 0,1 punti punti percentuali nel 2020. Anche le maggiori risorse per gli investimenti pubblici stanziate dalla legge di bilancio 2019 dovrebbero fornire un ulteriore stimolo alla domanda. Nel nuovo quadro tendenziale dei conti della pubblica amministrazione, gli investimenti aumenterebbero del 5,2 per cento nel 2019, già a partire dal secondo trimestre dell'anno, con un contributo alla crescita del PIL reale superiore di di 0,1 punti percentuali. Nel quadro programmatico dell'economia, che sconta gli interventi al varo (tra cui il cosiddetto sblocca cantieri), viene prudenzialmente stimata una crescita aggiuntiva dello 0,1 per cento (punti percentuali del PIL reale) nel 2019, che porta la crescita del PIL nello scenario ipotizzato allo 0,2 per cento in termini reali, rispetto allo 0,1 dello scenario tendenziale. Il Documento in esame reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede un incremento del PIL in termini reali e non nominali pari allo 0,2 per cento per il 2019 e allo 0,8 per cento per ciascuno degli anni 2020-2022. Il precedente quadro programmatico prevedeva un tasso pari all'1

Il precedente quadro programmatico prevedeva un tasso pari al 10,3 per cento per il 2019, con una successiva graduale riduzione fino a un valore pari al 9,4 nel 2021.

In un contesto economico congiunturale profondamente cambiato in peggio e, perciò, più complesso con questo Documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: la riduzione progressiva del *gap* di crescita con la media europea che ha caratterizzato l'economia italiana, soprattutto nell'ultimo decennio e, al tempo stesso, la riduzione del rapporto debito/PIL. Il conto economico tendenziale evidenzia per il 2019 e, in termini assoluti, pari a 42,1 miliardi. Per gli anni successivi il Governo stima, dunque, un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2019 sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL,

Il Governo intende, altresì, perseguire con il massimo rigore l'obiettivo della progressiva riduzione del rapporto debito/PIL, pur nel complicato scenario economico in atto.

è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente. La crescita tendenziale è stata ridotta dello 0,1 per cento per l'anno in corso a causa del riflettersi di un contesto di debolezza economica internazionale,

Il relatore di minoranza, senatore Misiani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non Signor Presidente, possiamo riassumere questo Documento di economia e finanza in due parole: fallimento e impotenza. I numeri del DEF certificano il fallimento della politica economica del Governo. Il 27 settembre, quando è stata presentata la Nota di aggiornamento, prevedevate una crescita dell'1,5 per cento. Tre mesi dopo il Governo ha ridimensionato le sue previsioni all'1 per cento e oggi leggiamo nel DEF che la crescita tendenziale quest'anno sarà dello 0,1 per cento e quella programmatica dello 0,2. Non è crescita; è stagnazione. Dalla metà del 2018 l'Italia ha perso 116.000 posti di lavoro e nel 2019 l'Italia sarà ultima per crescita tra i 39 Paesi avanzati. Siamo l'anello debole dell'Europa.

secondo i numeri del Governo, il 132,6 per cento. È il *record* dal 1924 ed è una stima ottimistica perché incorpora privatizzazioni per un punto di PIL che non verranno mai fatte. Peggiora la disoccupazione: doveva attestarsi al 10,3 per cento e toccherà l'11 per cento. Certo, pesa la congiuntura internazionale su queste previsioni, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, il rallentamento della zona euro, la frenata della Germania; molto, però, è dovuto a fattori nazionali. Ce lo hanno spiegato la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio e tutte le forze economiche e sociali che abbiamo udito.

è accaduto perché è crollata la fiducia dei consumatori, delle imprese e dei risparmiatori nei confronti del nostro Paese e quando crolla la fiducia si bloccano gli investimenti, si rinviano gli acquisti di beni durevoli e si tirano i remi in barca, in attesa di tempi migliori. Il motivo principale del crollo della fiducia è dato dall'incertezza politica dai dubbi degli operatori economici sulle intenzioni di fondo del Governo e della maggioranza. Signor Presidente, lo *spread* è il termometro finanziario della crisi di fiducia nel nostro Paese. Prima delle elezioni era inferiore a 130 punti, nei momenti più tesi dello scontro con la Commissione europea ha superato i 300 punti e da settimane è stabilmente superiore a 250 punti. Si tratta di una vera e propria stretta monetaria, che ci siamo autoimposti e che sta costando carissima al nostro Paese,

6 miliardi di euro in più nel 2021 e che ci sta costando cara in termini di mancata crescita, con una riduzione di 0,7 punti nel triennio, sempre secondo la Banca d'Italia. Badate che questa situazione è figlia di una politica economica sbagliata e di una legge di bilancio, che ha concentrato tutte le risorse disponibili su due misure quota 100 e reddito di cittadinanza - che costeranno 44 miliardi di euro in tre anni e 125 miliardi di euro in dieci anni. Sono due interventi finanziati in *deficit*, sottoscrivendo a nome di tutti gli italiani la maxicambiale degli aumenti IVA dal 2020 in avanti. Intendiamoci: rafforzare le misure contro la povertà era necessario in questo Paese e lo si poteva fare potenziando quello che c'era, ovvero il reddito di inclusione, evitando di ripartire da zero, ma avete fatto una scelta diversa. Ampliare i margini di flessibilità del sistema pensionistico era sicuramente opportuno. Lo si doveva fare in modo strutturale, però, non per tre anni, magari spendendo meno, ma concentrando le risorse sulle categorie più fragili e sui lavori usuranti, introducendo una pensione di garanzia per i giovani, andando avanti sulla strada avviata dal precedente Governo. Avete fatto le vostre scelte, avete impegnato soldi che il Paese non aveva e avete caricato di debiti le generazioni future. Lo avete fatto, sapendo che non ce lo potevamo permettere e azzerando ogni margine di manovra per le politiche di sviluppo. Avete guardato al presente, alle prossime elezioni, ma così facendo avete drasticamente ridotto i margini di intervento per il futuro. La vostra legge di bilancio ha ridotto le risorse per gli investimenti pubblici, ha smantellato gli incentivi per gli investimenti privati, ha aumentato la pressione fiscale sulle imprese. Avete bloccato i grandi progetti infrastrutturali, avete archiviato la revisione della spesa e non avete messo un euro in più sulla scuola e sulla ricerca. Non avete messo soldi sul futuro, ma avete badato soltanto alle immediate scadenze elettorali. Questi errori li stiamo pagando oggi,

e sono previsti in peggioramento i conti pubblici, con stime - lo ripeto - che sono peraltro ottimistiche, perché incorporano privatizzazioni che non farete

perché il Governo non ha una strategia, non ha una visione di politica economica e non ha un orizzonte temporale che vada al di là delle prossime elezioni europee. Vi siete chiusi in una dimensione di campagna elettorale permanente, ma così facendo avete rinunciato ad ogni ambizione di promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. E sull'ambiente, il vostro DEF, che incorpora un piano energia e clima ben poco ambizioso, gioca al ribasso; gioca al ribasso; Lo fa sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, sulle fonti rinnovabili, sullo sviluppo dell'energia solare e soprattutto non mette soldi ma poi taglia 300 milioni di euro al trasporto pubblico locale, mettendo a rischio un servizio essenziale per i cittadini e andando nella direzione esattamente opposta a quella dello sviluppo e della mobilità sostenibile che pure declamate nel DEF. Questa è la situazione, signor Presidente. Il Governo non ha una politica economica e non ha la più pallida idea di come impostare la manovra di bilancio del 2020. L'UPB ha fatto due conti sui soldi che servono: 25 miliardi nel 2020, 36 nel 2021 e 45 nel 2022 solo per lasciare le cose come stanno. Sono 106 miliardi in tre anni che dovete trovare l'Everest con le mani legate dietro la schiena ed è questa difficoltà che spiega la scelta del ministro Tria nel DEF di confermare l'aumento dell'IVA previsto dalla legislazione vigente. Quello che avete scritto, infatti, non è una mera formula lessicale. Nel DEF 2017 - l'ultimo programmatico dei Governi del centrosinistra - noi avevamo scritto delle cose chiare; avevamo scritto nero su bianco: «si prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia».

(a pagina 7, a pagina 39 e a pagina 48). Chi ha orecchie per intendere intenda, signor Presidente. Queste parole vogliono dire un'operazione verità (meglio tardi che mai): vogliono dire che l'IVA aumenterà fino a prova contraria, fino alla definizione di misure alternative che il vostro Governo non ha la più pallida idea di come definire. Questo è il punto che è emerso nel audizione del ministro Tria. anche una seconda certezza, al di là delle chiacchiere dei due Vice *Premier:* il taglio da subito di due miliardi di euro che avevate accantonato nella legge di bilancio. Lì dentro, signor Presidente, ci sono i 300 milioni di euro per il trasporto pubblico, ma ci sono anche 100 milioni di euro per l'università, per il diritto allo studio e per la ricerca, che tagliate subito, al di là dei proclami del Documento di economia e finanza. È inammissibile che questo Governo da una parte discuta di come ridurre le tasse a chi sta meglio con la *flat tax* e poi tagli i fondi per il trasporto pubblico e progetti di aumentare l'IVA. Questa è la cifra di fondo del Documento di economia e finanza: la reticenza, la rinuncia e l'attendismo nell'attesa di improbabili tempi migliori. Bisogna cambiare rotta, signor Presidente, e noi nella nostra risoluzione indichiamo alcune proposte nell'immediato e nel medio termine. Proponiamo di fare chiarezza sull'IVA (no all'aumento dell'IVA senza se e senza ma, perché è una misura depressiva e regressiva che colpisce il ceto medio e i ceti più deboli), di rimettere il debito pubblico su un sentiero discendente (altrimenti rischiamo grosso), spendere le risorse già stanziate (220 miliardi) per gli investimenti pubblici. Proponiamo inoltre, nel medio periodo, di trovare risorse per la scuola, per la sanità, per le urgenze vere di questo Paese, per il taglio del cuneo fiscale, facendo quello che finora non avete fatto: la revisione della spesa, le agevolazioni fiscali, i sussidi ambientalmente dannosi. Lo dico nel giorno in cui Greta Thunberg ha parlato al Senato della Repubblica: con sedici miliardi di euro noi finanziamo le fonti fossili, che danneggiano il clima del nostro pianeta e che voi non avete ancora avuto il coraggio di tagliare. Noi vi proponiamo di intervenire su questi punti e ci auguriamo che su di essi il Senato possa discutere con un dibattito costruttivo,

siamo in una situazione un po' strana, nel senso che si sta parlando di tre DEF: quello presentato dal ministro Tria, per il quale abbiamo fatto delle audizioni, e altri due dei quali si annuncia l'uscita, uno del vice presidente Salvini e l'altro del vice presidente Di Maio. Per il momento atteniamoci all'unico che abbiamo letto, perché degli altri due abbiamo visto solo dichiarazioni alla stampa.

che di politica economico-finanziaria del nostro Paese. Quest'anno c'è un documento che riporta un po' sulla terra le ambizioni di questo Governo.

da applicare sempre quando vanno su un terreno di gioco: è la regola del cosiddetto buon senso. Mi riferisco cioè a quell'atteggiamento complessivo che obbliga i giovani arbitri a usare un po' di intelligenza e di strategia per evitare situazioni spiacevoli.

Dove troviamo i soldi? Signor Vice Ministro, io la conosco e la apprezzo per il suo equilibrio e anche per la sua conoscenza tecnica, ma dove troviamo i soldi? Dei due decreti-legge di cui si parla moltissimo in questi giorni (quello sulla crescita e lo sblocca-cantieri) addirittura

Capite che sembra quasi un gioco fideistico quello di considerare questi dati taumaturgici di bellezza. Ogni tanto Ogni tanto mi piace ascoltare il presidente Bagnai che ci fa delle dotte dissertazioni e chiaramente io sono molto attento a quello che ci dice. Se dovessi collocare questo questo atteggiamento della maggioranza dentro i gironi danteschi, io li collocherei nell'ottava bolgia, laddove sono posti gli ingannatori e i falsi consiglieri

occorre un'operazione verità, dobbiamo dire agli italiani dove andiamo a trovare le risorse per sostenere queste politiche.

e i due Vice Presidenti del Consiglio. La borsa oggi non vi crede, non si fida e la mancanza di fiducia è il principale motivo per il quale la nostra economia non cresce. vengo dal Nord e anche al Nord si avvertono situazioni di disagio. Avevate citato, come unico dato positivo l'aumento della produzione industriale del mese di febbraio, tranne che stamattina l'Istat ha dichiarato che sono dati falsi. La produzione industriale a febbraio non è assolutamente cresciuta. Quindi, a maggior ragione, tutti quei dati di tendenza che sono stati individuati sono dati che dovrebbero imporre buon senso e prudenza. Lo sappiamo tutti: fra quindici giorni c'è una tornata elettorale, e sicuramente bisognerà raccontare agli italiani qualche balla, qualche frottola, perché non possiamo assolutamente sperare che ci sia un Ministro così competente come Tria mandato allo sbaraglio per poi, subito dopo, contraddirlo in maniera evidente. Tra IVA e privatizzazioni illusorie, avremo una manovra da sessanta miliardi senza sviluppo e con tre bilanci dello Stato a rischio. Ci sono delle riflessioni di fondo da fare. La prima è la non coerenza dei quadri macroeconomici con i conseguenti quadri di finanza pubblica. La seconda è la misura degli effetti delle politiche economiche del Governo espressa direttamente dal Governo. Il quadro di finanza pubblica indica un tasso di crescita del PIL per il 2019 pari allo 0,2 per cento, che balza dallo 0,2 allo 0,8 nel 2020, 2021 e 2022.

Di fatto, si tornerebbe nel 2021 ai tassi di disoccupazione annuali. Quindi, l'impatto e l'effetto delle vostre politiche economiche sull'occupazione è pari a zero: per tre anni non cresce

Si elimina, in questa maniera (ecco la dose di realismo che io riconosco al DEF), il miglioramento concordato prima di Natale nel famoso balletto che è stato svolto da questo Governo con la Commissione europea.

Si tratterebbe di una riduzione del 3,3 per cento in quattro anni, pari allo 0,8 per cento all'anno. Questi quadri macroeconomici risultano del tutto incoerenti con quelli di finanza pubblica. Il nodo consiste nel fatto che delle due l'una: se aumenta l'IVA, come previsto a legislazione vigente dalle clausole di salvaguardia, la crescita del 2020 andrà ben sotto lo zero, tra il -1 e il -2 se non aumenta l'IVA nel 2020, una crescita allo 0,8 per cento potrebbe anche essere raggiungibile ma, contestualmente, il *deficit* pubblico balza verso il 3,5 per cento e il debito pubblico andrebbe verso il 135 per riguarda gli effetti di politica economica. Gli effetti di politica economica che il Governo, non l'opposizione ma il Governo, si attende dalle sue politiche economiche

detto il Governo non noi. A fronte di questo minuscolo ed effimero impatto sulla crescita, la politica economica del Governo peggiora le condizioni di *deficit* e debito pubblico.

Le proposte di risoluzione relative al Documento in esame dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Ogni dichiarazione fatta prima di colazione in modo incauto provoca un danno di 2,4 miliardi di euro. Come ho già detto altre volte, dobbiamo stare attenti. Gli NPL nel sistema bancario sono indigeribili a queste dosi di Europa e, quindi, le banche stringono la borsa. Le dismissioni che avete previsto quest'anno sono pari a 17,8 miliardi di euro.

po'. Ci sono poi delle situazioni di difficoltà oggettiva. Il federalismo, se vogliamo dirla tutta in italiano, non si farà mai perché è una questione di soldi. Vorrete mica dire che se la Lombardia ha un *surplus* di 10 miliardi (non so se la cifra è giusta) e dice di non volerli versare più o versarne verso solo 5, il resto dell'Italia è disposta ad accettarlo trasversalmente? Il federalismo non è attuabile se attuato in modo diverso e io sono federalista.

la *flat tax* per tutti ho letto un articolo interessante che diceva: per attuare la *flat tax* bisogna avere un fisco come quello americano: se sbagli vai in galera. La giustizia, adottando il modello Davigo, per cui non esistono innocenti ma solo colpevoli che l'hanno fatta franca, non credo sbroglierà le questioni. Mi avvio a concludere. Occorrerebbero delle misure *shock*, come ai tempi del Governo Berlusconi. La legge Tremonti non è più proponibile, è cambiato il mondo quindi non serve più, ma ci vorrebbe una diminuzione secca delle tasse per tutti;

Concludendo, non si può vivere di sondaggi. Vivendo di sondaggi si fatica e allora si fanno delle misure che non danno risultati e che sono soltanto pura immagine. Attacchiamo il debito pubblico altrimenti il debito pubblico attaccherà noi. Prima di dare la parola al senatore Nencini, vorrei cogliere l'occasione per formulare gli auguri di buon compleanno al senatore Calderoli. Immagino che vorrà festeggiare questa sera con tutti i senatori a cena. *(Ilarità).*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le due relazioni di maggioranza e mi sono stupito che in entrambe le conclusioni entrambi i relatori abbiano sostenuto letteralmente: «Il Governo conferma gli obiettivi previsti». Non so a quali obiettivi ci si riferisca, perché - è già stato ricordato dal senatore Misiani - a settembre il Governo prevedeva una crescita dell'1,5 oggi ragioniamo su termini decisamente inferiori. Quindi abbiamo la certezza che la legge di bilancio approvata in maniera pirotecnica nel dicembre scorso debba essere completamente rivista.

Manca una visione strategica dell'economia nazionale; siamo in assenza di una collocazione dell'Italia dentro un quadro geopolitico profondamente cambiato - devo dirlo - nei momenti in cui la storia si avvita lungo tornanti di cambiamento profondo, se non c'è una relazione tra geopolitica e scelte strutturali dell'economia, è difficile uscire da

I numeri significati, non coincidenti, segnalano, però, una fotografia di un Paese in grave difficoltà. Mi limito a sottolineare, invece, un aspetto. Era mia opinione, fino ad alcuni giorni fa, che il Governo si muovesse secondo una logica da campagna elettorale permanente, come è stato detto; la logica che vedevo prevalente era quella di un presentismo continuo. Letto il Documento di economia e finanza, deve correggere anche questa opinione: non solo non si vede quale cornice strategica il Governo abbia a riferimento, ma io non leggo nemmeno quali siano i provvedimenti legati a un presentismo da campagna elettorale permanente. Cito i casi, uno per uno, traendoli dal Documento di economia e finanza (quindi non sono, Vice Ministro, opinioni personali). Non si parla di *flat tax* corredandola con numeri; si parla di aumento dell'IVA (perlomeno nelle dichiarazioni del Ministro che ha competenza piena sul tema); non esiste un piano di investimenti per le infrastrutture. Questa valutazione è stata oggetto anche di commenti e di un dibattito surreale all'interno dell'8a Commissione. allora, citare i documenti che sono stati prodotti dal Governo. Cito il titolo del capitolo: «Infrastrutture»; leggo: «Pur risultando assente, rispetto ai DEF precedenti, uno specifico Allegato infrastrutture (...), nel PNR riveste un particolare rilievo il tema del rilancio delle infrastrutture». Cerco, scavo, scartabello nel Documento di economia e finanza e non trovo una citazione né di un'opera da portare a conclusione, né di un euro da mettere per per fronteggiare la realizzazione di quell'opera. Quindi le dichiarazioni contenute all'interno del DEF sono assolutamente infondate. Vorrei essere, Vice Ministro, felicemente contraddetto, magari con numeri e con la citazione di un'opera che non sia generica, esattamente come il paragrafo che ho letto.

quindi corrispondente a verità ‑ mi rivolgo ai due relatori di maggioranza ‑ che il rapporto debito‑PIL stia diminuendo. È esattamente il contrario: il rapporto debito‑PIL aumenta, eccome se aumenta: è stato censito che è tutt'oggi, alle ore 16, più o meno in aumento, così come lo *spread*. *spread*. Signor Presidente, se un Documento così significativo per un Paese così significativo deve essere inserito all'interno di un quadro geopolitico, il Governo dovrebbe rispondere intanto su due questioni. La prima: cosa pensiamo dell'Unione europea? Perché una cosa è cambiarla, altra cosa è bombardarla quotidianamente. La seconda: se il *memorandum* che il Governo ha predisposto e siglato riguardante la Via della Seta abbia un significato di modifica del nostro assetto dentro le relazioni internazionali tipiche, quadro, di questo Paese. Concludo con un'opinione, che è naturalmente l'opinione personale di chi parla. Se non c'è strategia e se non c'è presentismo legato a una campagna elettorale imminente,

Giuseppe De Rita (che io chiamo ancora maestro), ritiene essere quella dell'uomo solo al comando. Non c'è altra scelta. scelta. Non prepariamo quindi con il Governo Conte alcuna scelta concreta per l'immediato: prepariamo una campagna elettorale e affidiamo ad un Governo balneare quale che sia - se non ad una campagna elettorale per le elezioni politiche, la soluzione finale per la Repubblica Italiana. È la ragione per la quale non parteciperò al voto.

il Documento di economia e finanza 2019 è il primo del Governo del cambiamento e fa seguito al programma di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento al DEF dello scorso autunno, poi concretizzatosi nella legge di bilancio. È vero, il documento rivede al ribasso il tasso di crescita del PIL italiano che però, nei primi mesi dell'anno, ha dato già qualche lieve segnale di ripresa, così come è emerso dalle proiezioni presentate qui in Parlamento, tra gli altri dall'Istat e dalla Banca d'Italia, in sede di audizioni sul DEF. La revisione delle stime di crescita va inserita in un contesto di rallentamento economico che, in dinamiche mondiali sempre più interdipendenti e interconnesse, deriva in buona parte dalle tensioni commerciali e dalle fibrillazioni legate alla Brexit. È di tutta evidenza, però, che ci troviamo in un momento di difficoltà peculiare dell'eurozona, all'interno del quale colpisce il rallentamento della Germania che ha sempre avuto una funzione trainante dell'economia europea. Il rallentamento sta colpendo il manifatturiero, un settore importante e caratterizzante dell'economia, sia tedesca che italiana. L'Italia, inoltre, risente di alcune condizioni di partenza sfavorevoli, come il differenziale di occupazione giovanile e femminile rispetto alla media europea; a questo si aggiunge un marcato calo demografico. Di fronte all'attuale contesto di fragilità economica, sia nazionale che internazionale, però, il Governo del cambiamento reagisce con responsabilità e con ancora maggiore convinzione, dopo aver approvato una manovra espansiva in controtendenza rispetto a tutte le manovre degli ultimi dieci anni, che puntavano soprattutto sui tagli e sull'austerità, manovre che non hanno mai condotto l'Italia ad una rinascita economica. Questo DEF delinea riforme espansive strutturali e organiche che intendono raggiungere risultati concreti e durevoli, grazie all'aumento del reddito disponibile delle famiglie, soprattutto di quelle meno abbienti, al sostegno ai consumi, al lavoro, agli investimenti innescati dalle misure contenute, in particolare, nei decreti crescita e sblocca cantieri in fase di finalizzazione. Il dato della crescita previsto nel DEF va anche inteso come molto prudenziale, considerando l'effetto sinergico delle numerose azioni che spingono nella medesima direzione ed è ragionevole pensare ad una crescita che possa rivelarsi superiore alle stime prudenti contenuta nel Documento. Il Governo e la maggioranza che lo sostiene intendono infatti agire su più fronti. Molte attenzioni sono dedicate alle piccole e medie imprese, autentica impalcatura del sistema economico. In questa direzione vanno letti gli interventi di alleggerimento del fisco, di semplificazione amministrativa e di tutela delle imprese in crisi. Per dare maggiore forza a queste politiche intervengono misure dirette a migliorare anche il contesto nel quale le imprese operano. Tra queste, molto opportunamente il Governo indica come prioritarie quelle che puntano alla tutela del *made in Italy*, alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, al rafforzamento del *venture capital* e del Piano impresa 4.0, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, alla promozione dell'innovazione tecnologica, essendo di vitale importanza per il Paese superare il *gap* sul digitale e affrontare la sfida del futuro che vede il veloce e inarrestabile processo di cambiamento in corso in tutti i settori. richiamato dal DEF, ci sono misure che disciplinano il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il rientro dei cosiddetti cervelli in fuga, cioè di quei professionisti - molti dei quali giovani - che per mancanza di opportunità sono stati costretti ad abbandonare i loro territori. Una misura tutt'altro tutt'altro che secondaria se si considera che il Fondo monetario internazionale registra per l'Italia il dato più alto negli ultimi cinquant'anni di giovani che fuggono all'estero. cambi di rotta necessari nei quali il Governo si sta impegnando, che sarebbero stati davvero utili anche negli scorsi decenni. Difatti, nello sblocca-cantieri - altro decreto richiamato dal DEF - si punta sulla ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione attualmente troppo ingessata

che territoriali. A questo si aggiunge l'importante piano contro il dissesto idrogeologico; un piano che incanala risorse stanziate nella manovra che finalmente dà priorità alla prevenzione. Il MoVimento 5 Stelle si è battuto fortemente per dare vita da subito al programma del reddito di cittadinanza, come sappiamo, con le sue basilari funzioni di sostegno al reddito e lotta alla povertà: strategia che allo stesso tempo intende rifondare le politiche attive sul lavoro. I risultati di questa complessa azione politica saranno visibili nei prossimi mesi perché realisticamente occorrerà un periodo di tempo congruo per raccogliere appieno i frutti e, in compenso, conseguiremo risultati di crescita stabile e duratura. Dovrei dire tanto altro. Certamente non ho detto tutto né avrei potuto in questi pochi minuti, ma, nel concludere, voglio ribadire l'impegno fermo del MoVimento 5 Stelle a non permettere alcun aumento dell'IVA. *(Applausi dai Gruppi M5S

sia sulle famiglie sia sulle imprese, stimolando investimenti e occupazione. Serve, signori, una seria e forte volontà politica. Nel Governo e nel MoVimento 5 Stelle questa volontà c'è; mi auguro che la medesima volontà affiori il più possibile fra tutte le forze politiche nell'interesse del Paese. Auspico, quindi, signor Presidente, la più ampia approvazione, da parte di questa Assemblea, del Documento di economia e finanza 2019.

FdI)*. Signor Presidente, mi accingo a discutere di questo Documento di programmazione economica e finanziaria con con l'animo di chi ha come bene primario l'interesse generale del Paese, e in questa ottica e con questa logica, l'atto al nostro esame presenta gravissime lacune, come tra l'altro hanno anticipato anche i miei colleghi di minoranza prima di me. Dopo alcuni giorni in cui abbiamo analizzato il testo in Commissione e lo abbiamo approfondito, anche alla luce delle numerose audizioni tecniche che si sono svolte alla presenza di illustri personalità della scena economica italiana, è venuto il momento di lasciare spazio alla politica. Questo Documento di economia e finanza, così come predisposto dal Governo di Lega e 5 Stelle, non può trovare assolutamente il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia. Perché dico questo? Perché, come emerso dall'analisi in Commissione bilancio, non vi è assolutamente una previsione di crescita,

Se fosse applicata, rappresenterebbe una vera boccata d'ossigeno per le famiglie e le nostre imprese: solo riducendo le tasse, infatti, possiamo sperare di far ripartire la crescita e i consumi. la *flat tax* era un tema condiviso dal centrodestra nella scorsa campagna elettorale e sarebbe dovuta rientrare tra i punti del programma di Governo. Questo DEF conferma invece che su tale assetto, strategico per l'economia del Paese,

il tradimento di una promessa elettorale in nome di un contratto di Governo che non sta portando da alcuna parte e che questo Documento dimostra essere praticamente insufficiente. Fratelli d'Italia si aspettava l'introduzione della *flat tax*, quella vera: in questo senso il nostro partito, con Giorgia Meloni, ha avanzato decine di proposte, tutte bocciate. Con questa premessa, abbiamo ragione di credere e di pensare che la linea economica dell'Esecutivo sia fatta da più tasse e burocrazia, ma poco sostegno a chi lavora e produce. Come Gruppo parlamentare non possiamo che essere delusi e preoccupati per la mancanza di certezze sul rischio dell'aumento dell'IVA, che - come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto - si evince in modo chiaro da questo Documento. Cosa comporta tale rischio? Le stime dell'Istat, istituto che abbiamo audito in Commissione e che certamente non è di parte, rivelano che un aumento dell'IVA porterebbe ad una contrazione dei consumi, ma soprattutto ad un aumento dei prezzi. Nello specifico, ha sottolineato come, con un aumento dell'IVA di 3,2 punti per l'aliquota ordinaria e di 3 per quella ridotta, l'effetto sui prezzi sarebbe maggiore di 2 punti percentuali nei mesi e negli anni successivi. L'aumento dell'IVA, dunque, non può prescindere da quello dei prezzi e sappiamo bene come questi aumenti si ripercuotano sulle fasce più deboli del popolo italiano. Dopo anni di crisi economica, in cui gli italiani hanno aggredito anche i loro risparmi, l'aumento dell'IVA si tradurrebbe in un ulteriore aggravio di spesa per i cittadini e le imprese. Capiamo che il Governo conti sulle misure assistenziali, come il reddito di cittadinanza, per la ripresa dei consumi, ma, purtroppo per l'Esecutivo, non è così che può funzionare: l'aumento dei prezzi infatti scoraggia i consumi, indipendentemente dai redditi che si andranno a percepire. La verità che vuole constatare è che questo Governo, sull'aumento dell'IVA, stenta ad assumere una posizione chiara, preferendo invece puntare tutto sull'assistenzialismo del reddito di cittadinanza, quando invece sarebbe opportuno frenare e scongiurare l'aumento delle tasse e delle imposte.

bene, trovi lei le alternative, lei è Ministro della Repubblica ed è lei che ha il compito di trovare la soluzione a questo problema, che porterebbe l'Italia in una recessione devastante. Vi è anche un altro rischio concreto: che aumentino le imposte e le tasse e non si riduca il debito. Questo è quello che dice il Documento di programmazione economica Il quadro previsionale su cui si sta lavorando produrrà un ulteriore aumento del debito pubblico, senza alcun affetto sulla crescita, creando un paradosso: più debito, meno crescita. Non migliorano i conti e non migliorano le condizioni di vita degli italiani, che anzi rischiano di trovarsi letteralmente appiedati. Perché dico questo?

all'interno del Fondo nazionale dei trasporti, da cui vengono detratti questi 300 milioni di euro. L'allarme è stato lanciato dalla Conferenza delle Regioni, per tramite dell'assessore al bilancio della Regione Lombardia e l'appello fatto da questo assessore non può rimanere inascoltato. A dicembre - come è stato riferito in Commissione - si rischia che i mezzi per il trasporto pubblico locale rimangano nei depositi; c'è il pericolo concreto che gli enti locali si ritrovino nell'impossibilità di rispettare i contratti sottoscritti con le aziende di trasporto locale e i tempi di pagamento ai propri fornitori. Questo ulteriore taglio da 300 milioni di euro è un provvedimento che va anche contro gli obiettivi ambientali e fa il paio con il rifiuto di alcune infrastrutture, come l'Alta velocità Torino-Lione, che sono invece strategiche per una nuova cultura della mobilità legata alle ferrovie, che sono il sistema di trasporto meno impattante per il nostro ambiente. ambiente. Noi di Fratelli d'Italia auspichiamo l'apertura dei cantieri per le grandi opere, che frutterebbero oltre 150.000 posti di lavoro. *tax*. Questa è la ricetta che avremmo voluto leggere nel Documento che stiamo ora discutendo. Inoltre, non c'è traccia di crescita neppure per i nostri giovani. Anzi, il DEF prevede una riduzione delle spese per sostenere l'istruzione, che passano al 3,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2021, per poi scendere ancora di più negli anni successivi. Diminuiscono quindi le spese per la scuola e per l'università. Se queste sono le scuole che vogliamo dare ai nostri figli, poi non ci lamentiamo se preferiscono andare a studiare e a lavorare all'estero. Questa è la prova provata che non state investendo sul futuro dei nostri figli. Inoltre, in questo DEF Fratelli d'Italia non vede prospettive e non vede investimenti, ma solo appunti sulla spesa corrente. Quello che emerge, in definitiva, è che tutto è rimandato: la crescita è rimandata, la possibilità di scongiurare l'aumento dell'IVA è rimandata, la *flat tax* è rimandata, un po' come se fossimo a scuola. Permettetemi di dire che anche il Governo è rimandato, perché preferisce mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che agire. L'imperativo è aspettare; del resto, siamo in campagna elettorale, le scelte coraggiose sono anche scelte rischiose, e allora è chiaro che avete preferito aspettare il 26 maggio, come se non ci fosse un domani dopo le elezioni europee. Fratelli d'Italia prende atto di un DEF inconsistente per questo Parlamento e per la nostra economia nazionale. Inoltre oggi noi presentiamo all'Aula una nostra proposta di risoluzione, che prevede punti ben precisi; tra gli altri, l'eliminazione della clausola di salvaguardia che prevede l'aumento dell'IVA,

dentro il quadro macroeconomico contenuto nel Documento di programmazione. Tutte le stime del Fondo monetario, dei principali centri studi e delle autorità indipendenti mostrano una generale revisione al ribasso delle prospettive di crescita per i Paesi più avanzati, ancora più consistente in Europa. Il tutto avviene all'interno di un quadro di profondi e rapidi mutamenti dell'andamento del commercio mondiale. Scenari che sono recepiti nel DEF, il primo vostro DEF, che necessariamente deve consolidare, nei saldi di finanza pubblica e nel PIL tendenziale, gli effetti e le ricadute della legge di bilancio e dei principali provvedimenti del contratto di Governo tra Lega e 5 Stelle. Diciamo subito, onorevoli senatori, che questa cornice macroeconomica viene recepita in ritardo, in quanto era già prevedibile con la legge di bilancio. Potremmo dire: meglio tardi che mai, benvenuti nella realtà e soprattutto consapevoli che siete al Governo del Paese. Non era difficile prevedere in anticipo le misure necessarie per sostenere la crescita e lo sviluppo. Bastava ascoltare tante proposte, alcune anche da noi avanzate. Bastava ascoltare con maggiore attenzione l'analisi delle autorità indipendenti, delle parti sociali e delle associazioni economiche, che sin dalla fine del 2018 indicavano questo quadro macroeconomico. Con altrettanta chiarezza e nettezza, riteniamo che, proprio all'interno di questo quadro macroeconomico, si consumi il vostro fallimento. Il DEF, inadeguato, senza spina dorsale, tutto piegato e orientato a generare aspettative per la campagna elettorale che pare non esaurirsi mai, produce incertezze gravi e pesanti a carico dell'economia, delle famiglie e delle imprese di questo Paese. Se teniamo insieme questo contesto con la propensione che fin qui avete sviluppato del fare opposizione al passato, i danni che state producendo rischiano di essere costosi per i giovani innanzitutto, per l'Italia che produce e lavora, per le famiglie e per le imprese che - non dimentichiamolo mai - sono il cuore di una comunità. Il DEF è un'occasione mancata: non individua un progetto; non indica una priorità. Esaurisce, a mio avviso, il ciclo positivo che avete generato con le elezioni, che avete consumato rapidamente all'interno di una mediazione impossibile di due progetti competitivi (quello della Lega e quello del MoVimento 5 Stelle) che via via hanno assunto maggiore distanza e maggiore competitività. Insieme diventano insostenibili e, quando sono insieme, spesso sono alternativi e competitivi e producono danni culturali e ideologici molto rilevanti nel nostro Paese. Le misure introdotte con la vostra legge di bilancio consolidano nel bilancio della pubblica amministrazione un dato preoccupante che, a nostro avviso, rischia di parcheggiare l'Italia in recessione per molto tempo. Il collega Misiani ha già indicato con chiarezza, nei numeri e nei dati, questo quadro e questo contesto. Basta leggere le relazioni della Banca d'Italia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Emerge con chiarezza un dato strutturale molto preoccupante: nel 2018 le spese sono cresciute dell'1,2 per cento meno del prodotto e di 9,3 miliardi di euro nel complesso.

Se a questo aggiungiamo le ricadute delle scelte politiche più importanti che hanno manifestato esiti non propensi allo sviluppo e alla crescita - mi riferisco al reddito di cittadinanza e a quota 100 nel 2019 si aggiungeranno altri 15,2 miliardi e 33 nel triennio, oltre 50 miliardi di euro di spesa sottratta al debito e agli investimenti. Questo è un quadro preoccupante e strutturale, che non presenta alcuna soluzione. Ecco perché il DEF consolida l'aumento dell'IVA. Rischiamo di essere il Paese con l'IVA più alta, con una conseguente regressione dei consumi e a pagare sono sempre le famiglie, proprio quelle meno abbienti, che si vedono ridurre ulteriormente il loro potere d'acquisto. La riduzione dell'occupazione e l'incremento della pressione fiscale che state generando e che si scaricherà nel 2019 attraverso anche uno sblocco di pressione fiscale, che oggi porta molti Comuni e molti territori a incrementare l'Irpef, l'IMU e la Tasi,

trimestri di crescita, abbiamo già attraversato due trimestri in recessione tecnica. Non ci voleva molto ad anticipare misure coerenti per la crescita e lo sviluppo. Lo state facendo con un ritardo enorme, con un'incomprensibile inadeguatezza, che diventa per certi aspetti una vergogna, perché stiamo discutendo di un Documento di programmazione economico-finanziaria che incorpora già misure che questo Parlamento non conosce relative alla crescita, allo sblocca cantieri e al rilancio degli investimenti. qualcosa di incomprensibile perché, dopo sei mesi di recessione tecnica, bastava anticipare queste misure per rendere più fluido e più coerente un'idea di sviluppo di questo Paese. questo Paese. Questo è il DEF. Purtroppo, è un DEF che nasconde tante promesse: sono i pagherò che mi preoccupano e che ci preoccupano. Vedete, sull'IVA si sta giocando sulla pelle degli italiani. Lo voglio dire ai colleghi del MoVimento 5 Stelle:

chiarezza, perché questo tipo di impostazione e soprattutto i pagherò scaricano sul debito e sulla spesa corrente oneri insostenibili. Avete costruito un'idea di *spending review* senza riforme e senza spina dorsale. Ricordiamo che, per evitare che la riduzione della spesa si scarichi su minori servizi pubblici e sulla scuola, e sulla scuola, abbiamo bisogno di invertire le tendenze. Oggi servirebbe un'unica misura per lo sviluppo e per rilanciare la crescita: un nuovo modello economico e sociale, che preveda la riconversione in chiave ecologica dell'economia. Occorrerebbe ridurre il cuneo fiscale, ridurre il costo del lavoro e aumentare i salari minimi per i lavoratori e le famiglie.

onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un DEF molto prudenziale e non potrebbe essere diversamente, perché in realtà si tratta di un documento che arriva adesso, in aprile, quando notoriamente gli effetti della legge di bilancio di dicembre non si possono ancora quantificare e le misure devono ancora entrare a regime. Facciamo però un po' di storia recente. Veniamo da anni di straordinaria congiuntura internazionale positiva, con il petrolio ai minimi, interessi ai minimi con il *quantitative easing* di Mario Draghi, un cambio tra euro e dollaro favorevole, eppure l'Italia è rimasta fanalino di coda. vorrei ricordare al collega Manca che abbiamo già disinnescato una volta la clausola di salvaguardia IVA e quindi bisognerebbe fare chiarezza su questo visti i risultati degli ultimi anni, con la legge di bilancio abbiamo voluto cambiare strategia rispetto al passato. L'esperienza dei Governi Monti, Renzi e Gentiloni Silveri insegna che a puntare sulla riduzione del *deficit* per ridurre il debito, con politiche restrittive, che penalizzano il PIL, si ottiene un risultato peggiorativo, con un debito che, nello specifico, è passato da Monti a Gentiloni Silveri, dal 120 per cento al 132 per cento del PIL: è evidente che le manovre di quei Governi non erano sulla strada giusta. *(Applausi e M5S).* Non pretendiamo di avere la bacchetta magica, ma almeno ci deve essere lasciata la possibilità di cambiare registro. La manovra di bilancio ha voluto agire sui fondamentali dell'economia italiana: domanda interna e investimenti. Lo ha fatto attraverso le misure cardine di quota 100 e del reddito di cittadinanza, stimate prudenzialmente nei loro effetti ancora da verificare, ma che sicuramente daranno impulso alla domanda delle categorie più deboli e ad una maggior vivacità del mercato del lavoro, con un indubbio ricambio generazionale. Anche la stima delle nuove assunzioni, a fronte dei pensionamenti in base alla cosiddetta quota 100, pari al 30 per cento, sembra essere troppo bassa e troppo prudenziale. misure di impulso alla domanda interna, sia per quanto riguarda gli investimenti pubblici, sia in termini di incentivi alle aziende. La grande sfida è quella di riuscire a rimettere in moto un Paese bloccato.

che all'opposizione sembrano forse di poco conto, ma che vanno ad agire e ad iniettare risorse subito spendibili sul nostro territorio, che è fatto di piccole e di microrealtà. nel settore privato, la mini *flat tax*, la tassazione al 15 per cento per ricavi fino a 65.000 euro, la tassazione del 5 per cento per le nuove partite IVA, la cedolare secca per i nuovi affitti commerciali, il raddoppiamento della deducibilità dell'IMU sui capannoni, la riduzione dei premi INAIL del 30 per cento, che va ad agevolare in particolare il settore edile delle costruzioni, la riduzione dell'IRES sugli utili reinvestiti: tutte misure per mettere pace tra fisco e contribuente, misure puntuali,

Così nella frammentazione delle realtà locali, come nella particolarità della composizione del tessuto aziendale italiano, per oltre il 95 per cento composto da piccole e microimprese. Certo, c'è ancora tanto da migliorare, tanto da fare. Sarà prossima quindi la pubblicazione del decreto crescita, in continuità con le politiche fin qui attuate, sulla scia dello stimolo della domanda interna e che va nel senso di agevolare ancora più il settore pubblico e privato. Il decreto sblocca cantieri, che va nella direzione della semplificazione e revisione di quel codice degli appalti complice del blocco degli investimenti pubblici in Italia. Tutte misure che vedranno i loro effetti, però, nei prossimi mesi. Ma intanto oggi, dopo la grave flessione dell'attività produttiva dovuta a fattori esogeni, manifestatasi in particolare nell'ultima parte del 2018, l'industria italiana ha registrato una netta ripresa nei primi due mesi del 2019. L'indice della produzione industriale ha registrato un incremento congiunturale dello 0,8 per cento, confermando i segnali positivi di gennaio cento e l'andamento recente della produzione industriale italiana mostra una maggiore vivacità rispetto sia a quello dell'area euro (-0,2 per cento a febbraio, +1,9 a gennaio), sia a quello della Germania (-0,2 a febbraio e -0,4 a gennaio), anche se il senatore Ferro dice che questi dati non sono giusti, ma io mi attengo a quelli che sono stati consegnati nelle audizioni. audizioni. Dopo questo DEF arriverà la NADEF a settembre, maggiormente supportata dai primi risultati reali per poi trovarci, a fine anno, in legge di bilancio, dove si potranno realmente tirare le somme del primo anno di politica economica di questo Governo. Ad oggi, l'emissione di un Documento di economia e finanza prudenziale è scelta corretta

Signor Presidente, Vice Ministro, colleghi, nel Documento economico-finanziario del 2018 avevo dichiarato, nella mia prima esperienza parlamentare, il mio dispiacere, come italiano, nel prendere atto della lontananza del DEF rispetto ai veri problemi del Paese. Oggi, che discutiamo del DEF del 2019, non solo sento un dispiacere maggiore rispetto ad allora, ma sento di dover affermare che state mettendo in atto verso gli italiani e verso il nostro Paese un vero e proprio *bluff* politico istituzionalizzato. Questo DEF, colleghi, è sostanzialmente inutile per il nostro Paese, perché è privo di contenuti reali. Dice poco sulla sanità, non vi è traccia sulla rendicontazione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, utile a comprendere se gli impegni di spesa vengono rispettati. Non vi è traccia delle grandi opere, della TAV, necessarie per rendere competitivo il nostro Paese e creare occupazione. L'unica certezza riportata virgolettata nel DEF è l'aumento delle accise dell'IVA che possono scattare dal 22 per Ad oggi, nel 2019, siamo costretti a prendere atto soltanto dei fallimenti economici e finanziari e delle vostre misure, dei vostri *spot.* La quota 100 sta provocando la fuga di molti dipendenti dagli enti locali e anche e soprattutto dalla sanità, già in ginocchio perché sotto organico e nel DEF non è previsto alcun aumento del Fondo sanitario per sbloccare il *turnover.* La *flat tax* è rivolta a una platea ridottissima, perché si rivolge soltanto a chi fattura meno di 65.000 euro. Cosa diciamo a tutti coloro che oggi non lavorano, a tutti quei medici, parlando di sanità? Sono oltre 30.000 gli specialisti, che hanno studiato più di 25 anni e che non hanno un lavoro: cosa diciamo loro, che non sblocchiamo il *turnover*? Fate la domanda per avere il reddito di cittadinanza? È questo ciò che propone il Governo? Oltretutto, il reddito di cittadinanza inizia a smascherare la propria natura: gli stessi cittadini postano sui *social* l'elemosina di Stato, i 20, 30, 40 euro di reddito ottenuti dopo che sono stati ammessi al al beneficio, cioè hanno avuto la triste sorpresa di apprendere che l'importo del sussidio è di poche decine di euro. Di sussidio, infatti, si tratta e non, come avete detto e stradetto, di una misura per abbattere la povertà: non si abbatte la povertà con questo reddito di cittadinanza! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Colleghi, il Paese ha bisogno che si affrontino i temi del lavoro, dell'impresa, del Sud, delle infrastrutture, della sanità, del *welfare,* ma in maniera seria e concreta.

perché avete creato un Ministero che, oltre a non avere il portafoglio, non ha prodotto alcun progetto di investimento al Sud. E ancora oggi venite a riunirvi, come Consiglio dei ministri, a Reggio Calabria, Calabria, ma per annunciare cosa? Che avete partorito il topolino dalla montagna, mentre la gente muore, perché non ha assistenza sanitaria e continuerà a non averla per il decreto-legge

assoluto della politica sanitaria nazionale. Per l'anno corrente ci preoccupa che per la spesa sanitaria si prevedano 118 miliardi di euro, un aumento di soli 2,5 miliardi rispetto all'anno precedente, quando nella legge di bilancio ne avete previsto soltanto uno: dove prendere il miliardo e mezzo che avete aggiunto? aggiunto? Per gli anni successivi ci preoccupano le revisioni al ribasso del PIL rispetto a quanto avete preventivato sei mesi fa,

la spesa sanitaria resti inferiore all'inflazione. Anche se le vostre stime fossero corrette, la spesa sanitaria non potrà nemmeno coprire l'aumento dei prezzi, sia perché cresce meno del PIL nominale, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale dei prezzi al consumo.

usare parte della spesa sanitaria, oggi destinata all'assistenza sanitaria, per pagare l'aumento dell'IVA e non le prestazioni che già mancano, come dimostrano le lunghe liste d'attesa. liste d'attesa. La vostra politica economica ci dice che se hai bisogno di curarti o hai i soldi o muori; che se vuoi avere un lavoro o vai all'estero o vieni mortificato da poche decine di euro; che se hai un'impresa o ipotechi tutto con le banche, sperando che il prossimo DEF preveda una vera e propria *flat tax,* oppure vendi la tua azienda per pagare i debiti. Questa è l'Italia che avete disegnato nel vostro DEF: se non siete in grado di affrontare i problemi chiave dell'Italia in maniera seria e concreta, lasciate il Governo, lasciateci liberi, lasciate liberi gli italiani. Signor Presidente, vago, inattendibile, inutile è il DEF che il Governo presenta. una provocazione e un'offesa, perché costringe il Parlamento a una discussione inutile, svuotandolo di senso e di ruolo; un atto di estrema gravità che denunciamo ancora una volta. Avremmo potuto scegliere di sottrarci a questa pantomima restando in silenzio, ma abbiamo troppo rispetto di quest'Aula e della democrazia parlamentare. DEF inutile ma, per i vuoti che determina e le questioni che apre, enormemente pericoloso, perché conferma, una volta di più, la totale inadeguatezza di questo Governo a fronteggiare la fragilità del Paese, avendo ereditato (lo dico in premessa, perché non voglio più ripeterlo), tutte le condizioni per agire in un'altra direzione e oggi ragionare su ben altri indicatori. Sui rischi si sono espressi con puntualità di analisi tutti quanti sono stati auditi nelle Commissioni bilancio. Non solo le parti sociali, ma anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei conti, Bankitalia e l'ottima relazione del nostro relatore, senatore Misiani. Potete fare spallucce quanto volete: questo DEF è la certificazione di un fallimento e, soprattutto, della totale assenza di pensiero e strategia su come si difende il nostro sistema-Paese e il suo ruolo in Europa e nel mondo. La priorità, come costruire lavoro e buona occupazione, voi l'avete messa sotto il tappeto. È il punto giù grave, non può essere taciuto. Altrimenti, il decreto crescita non sarebbe al palo e, in quest'Aula, ministri come Di Maio e Lezzi avrebbero saputo come rispondere quando gli chiedevamo che fine avessero fatto Industria 4.0, il credito di imposta per l'innovazione e la ricerca, le aree di crisi complesse, i tavoli di crisi, le misure per il Mezzogiorno da noi messe in campo e da voi cancellate. Non hanno risposto. Non sapete rispondere. Voi non avete cancellato la povertà, come è evidente, per la debolezza di attuazione che sta registrando anche il vostro reddito di cittadinanza: chi dovrà sostenere le persone nella ricerca di un lavoro non arriverà prima della fine dell'anno e sul sito dell'Inps avanza la disperazione di chi comprende che questo reddito non sarà quello che sperava. State distruggendo questo sistema-Paese, disorientando e indebolendo chi produce (regime dell'incertezza, così lo hanno definito gli osservatori) e allontanando scientemente gli investitori.

Avete smantellato politiche industriali e strategia per il Mezzogiorno. State, colpevolmente e consapevolmente, tagliando le gambe alla seconda manifattura europea e settima nel mondo.

da mesi in Germania discutono su un piano strategico industriale che punta in modo esplicito alla creazione di grandi campioni europei nei settori strategici dell'industria. La più grande manifattura europea, quella cui guardano le Regioni settentrionali che chiedono l'autonomia rafforzata, illudendosi che questa sia la soluzione, mentre è evidente che non lo è, si interroga su come rispondere alla crisi. Non fa balletti come i vostri, tra Tria e i Vice *Premier*, su IVA sì o IVA no. Non inventa strategie di distrazione di massa, come quella sulla legittima difesa da voi inscenata. *(Applausi dal Gruppo PD)*. No: si interroga con un grande dibattito pubblico su come sostenere le proprie imprese, difendere le proprie eccellenze, trattenere i propri giovani, parlare da pari a pari con i giganti mondiali. Pensa all'interesse nazionale, quello da voi sbandierato e quotidianamente smentito, come dimostrano i vergognosi andirivieni su cantieri, opere pubbliche, infrastrutture, inutili quanto sbagliate analisi costi-benefici. Mentre voi, per affossare ancora di più il Mezzogiorno, abolite la clausola del 34 per cento che noi avevamo indicato per legge. Sì, a parole la sostenete, di fatto, ampliarla a Ferrovie e ANAS, che con i nostri programmi già viaggiavano intorno al 43 per cento di risorse per i territori meridionali, equivale a vanificarla. E non vi assolverà un Consiglio dei ministri fatto a Reggio Calabria, vuoto di contenuti e di proposte! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Davanti a tutto questo voi ci presentate un documento vuoto e inattendibile. Più *deficit*, più crescita e meno debito: così Tria sintetizzava la strategia del Governo, rinnegando impegni passati e sottostimando il costo per il bilancio delle misure proposte. Questo DEF vi smentisce su tutta la linea; smentisce l'anno bellissimo di quel burlone del presidente del Consiglio Conte; smentisce il duo Salvini e Di Maio

Smentisce l'impatto atteso - solo da voi - dalle vostre misure bandiera su crescita e consumi. Le stime reali sono molto al di sotto delle soglie immaginate e, come vi avevamo spiegato, non saranno quei consumi a sostenere la produttività della nostra dorsale economica, né internazionalizzazione ed *export*, di cui vi state irresponsabilmente disinteressando. Il reddito di cittadinanza è ben sotto le attese. I giovani che lo hanno chiesto sono meno di 25.000, le famiglie numerose sono tagliate fuori e così gli indigenti. Di Maio esulta dicendo che avanzeranno i soldi. Che dire, se non: vergognoso? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quota 100 non determinerà un *turn over* in un quadro economico così critico. Lo sapete anche voi, perché avete ipotizzato un aumento minimo di posti di lavoro. State solo continuando a bruciare miliardi a *deficit* e aumentando ulteriormente il debito pubblico, da perfetti giocatori cinici e bari. Caro vice ministro Garavaglia mi ascolti, anche se non le fa piacere quello che dico, ma è un suo dovere ascoltarmi. State massacrando il Paese e il futuro dei ragazzi e delle ragazze. Per questo, noi diciamo no a questo documento e vi sfidiamo a una discussione vera - quella che non avete voluto fare nelle Commissioni, in quest'Aula e dovunque - su quello che veramente serve al Paese e su come si difende veramente l'interesse nazionale.

un contesto congiunturale economico in cui la crescita mondiale rallenta, principalmente per la riduzione del commercio globale, il nostro Paese ha tenuto. Segnali positivi arrivano dall'Istat per quel che riguarda la produzione industriale. Nell'ambito di una sana dialettica politica, noi parlamentari esprimiamo diversi punti di vista. Difficile stabilire chi ha torto o chi ha ragione. Sicuramente, come esponente della Lega facente parte della maggioranza, sono a difendere la linea tracciata da questo Governo. Vista la vastità della materia del Documento di economia e finanza, mi soffermerò solo su alcuni aspetti. Apprezzo che, secondo l'accordo di maggioranza contenuto nel contratto di Governo, si intenda procedere con la prossima legge di bilancio con il processo di riforma sui redditi (*flat tax*) e di semplificazione del sistema fiscale, andando incontro alle istanze del ceto medio. Porto solo un esempio dei molti apprezzamenti su quel che è già stato fatto finora, ricevuti da persone e piccoli imprenditori che tutti i giorni lavorano a testa bassa e che non chiedono altro che lavorare e non impiegare il loro tempo a rincorrere la burocrazia. Marta, una restauratrice di Verona, già ora, secondo le attuali regole della *flat tax* per i redditi sotto i 65.000 euro, dice che lei è contenta perché dal commercialista già ora ci dovrà andare una volta l'anno non ha più l'incombenza dell'IVA trimestrale. Anche se non potrà più detrarre le spese, ha i clienti che, non essendo più assoggettati all'IVA al 22 per cento, sono incentivati a spendere un po' di più e a rivolgersi a lei. L'unica incombenza sarà quella di usare una marca da bollo di 2 euro superando i 77 euro per fattura. Coloro che apriranno una partita IVA potranno, all'inizio, scegliere una riduzione INPS dai 900 ai 600 euro trimestrali, che ovviamente creerà loro iniziali lacune contributive, ma che permetterà all'inizio di avere meno bisogno di liquidità. Secondo lei, incrementando ancor di più il tetto dei 65.000, si incentiveranno quei giovani che, non trovando lavoro presso le aziende, potranno aprire una partita IVA. Altra importante questione è quella delle culle vuote, ossia il calo demografico. Nel DEF si intende proseguire nell'attuazione di politiche volte a invertire le tendenze demografiche avverse, nonché a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la natalità e la genitorialità. Il nostro intento politico è invertire questo *trend* venendo incontro alle esigenze delle famiglie secondo il motto «prima gli italiani». Certo, massimo rispetto e impegno per gli immigrati ben integrati e che rispettano le regole del nostro Paese, che li ha accolti. Certamente a differenza di prima e di altri, noi della Lega non cercheremo di compensare il calo demografico spalancando le porte e i porti italiani. Da sindaco di un Comune, ho sempre la speranza che le nostre comunità nel futuro brulichino di bimbe e bimbi e di vedere le aule scolastiche con un maggior numero di alunni. È mortificante per un sindaco vedere pochi alunni in classe. E se chiudono le scuole elementari dei piccoli Comuni, anche le municipalità perdono di senso. Significativo sarà che il nostro Paese torni ad essere uno degli attori principali nello scacchiere europeo, quindi sarà molto importante vedere come si esprimeranno gli elettori il prossimo 26 maggio. Tornando al DEF, il tempo e gli elettori diranno la loro. Siamo politici e giustamente e democraticamente gli italiani ci giudicheranno con il voto. Come succede per i sindaci, chi ben amministra viene riconfermato alla guida del proprio Comune. Chiudo il mio intervento, augurando una buona e santa Pasqua di Resurrezione ai dipendenti del Senato della Repubblica, ai dipendenti dei vari Gruppi legislativi, ai colleghi parlamentari, alla Presidenza del Senato e ai membri del Governo.

Presidente, colleghi, membri del Governo, il DEF 2019, il primo elaborato dal Governo in carica, ripercorre i risultati conseguiti nei primi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma per il prossimo triennio. Cari colleghi, scusate l'ironia, ma se i risultati conseguiti sono quelli sotto gli occhi di tutti gli italiani, c'è da essere veramente preoccupati. Questo Governo sta creando le migliori premesse per fare incubare dall'Italia la prossima crisi finanziaria internazionale: il bilancio italiano può far saltare l'economia mondiale e viene trattato secondo le modalità tipiche del populismo latino-americano. Questo DEF è un Documento dove si evidenziano plasticamente le contraddizioni di questa maggioranza, Lega e 5 Stelle. al DEF 2018, presentate ad ottobre, mancava una giustificazione alla proiezione di crescita per il 2019 dell'1,5

per i tre anni successivi; e non è chiaro, oggi come allora, come si possa realizzare un incremento dello 0,6 per cento in un anno tra il 2019 e il 2020. Non è specificato per quali ragioni, una volta raggiunto lo 0,8 per cento di crescita, questo dato si fermi. Il Governo giallo-verde continua a ricorrere alla spesa in *deficit*, non giustificata da una crescita del PIL, che è largamente inferiore ai tassi di interesse medi pagati sui nostri titoli di Stato. In poche parole, cari amici, questo Governo compra consenso con l'aumento della spesa pubblica prima delle elezioni europee. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un atto gravissimo, che abitua i nostri giovani a non far niente, fannulloni con le sovvenzioni dello Stato, mortificando meritocrazia, impegno, sacrificio: una vera e propria vergogna. Non si può fare continuamente campagna elettorale sulla pelle degli italiani e non è la prima volta che ve lo dico: fate orecchie da mercante. Basta! Smettetela di raccontare l'Italia come un Paese diviso tra un Sud che non vuole lavorare e un Nord che lavora, ma che non vuole pagare le tasse: è un'idiozia, che alimenta una frustrazione sociale tra le due aree del Paese. Non contenti, continuate con infinite promesse un *mix* di propaganda elettorale per il nostro Paese. Ve lo ripeto ancora: zero assoluto sulla scuola; zero assoluto sulla ricerca; zero sull'innovazione; zero per lo sviluppo del Mezzogiorno; il Sud, totalmente dimenticato e assente nel famoso contratto; zero sulla natalità; zero sull'occupazione femminile; zero per le donne con i figli; zero per la redistribuzione fiscale a favore dei giovani e tanto Il Governo - si legge nella relazione - ha poi intenzione di accrescere la competitività del Paese a livello internazionale. Ma come si come si fa a fare tale affermazione, quando negli ultimi dodici mesi avete fatto andare via dal nostro Paese 118 miliardi? Erano i soldi degli investitori italiani ed esteri messi su imprese e buoni del Tesoro. Cosa avremmo potuto fare con quei 118 miliardi? Quanti investimenti saremmo riusciti a fare, senza aumentare il debito pubblico? Fa venire la pelle d'oca il capitolo che parla di opere pubbliche e investimenti per le infrastrutture. Bloccate le grandi infrastrutture che collegano l'Italia al resto d'Europa; danneggiate soprattutto le Regioni meridionali - sì, il Meridione, come sempre - quelle maggiormente depresse e quindi più bisognose di interventi. Nel DEF si parla di "strategia Italia", ma è assolutamente evidente che nel Governo ci sono tre strategie: una di Tria, una di Di Maio e una di Toninelli. Auguri!

quello in cui i due Vice *Premier* non rivelano come hanno intenzione di realizzare la *flat tax* e soprattutto con quali coperture finanziarie; poi, il terzo DEF, tutto da ridere, quello di Toninelli, che nel bel mezzo di un'intervista televisiva fa finta di non conoscere quello approvato dal suo Governo. A quale delle tre versioni dobbiamo credere? Questa linea ondivaga è oramai intollerabile. Ci troviamo in uno scenario agghiacciante, che genera incertezza sui mercati e in Europa, che mette i bastoni tra le ruote alle imprese, incapace di fare un minimo di programmazione. facendo notare a tutti un fatto gravissimo: la scomparsa di ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania, denunciata proprio ieri dal capogruppo regionale di Forza Italia Armando Cesaro. *(Applausi dal ha il dovere di spiegare con assoluta chiarezza i motivi per i quali ha sottratto alle politiche economiche campane il 20 per cento dei circa 10 miliardi di euro destinati a programmi di sviluppo del lavoro, non ultimo quello di Fincantieri di Castellammare. Presidente, amici del Governo, il fatto che a tagliare le risorse alla Campania sia un Ministro del Sud, napoletano, di Pomigliano, rende questa vicenda ancora più grave, vergognosa, paradossale.

onorevoli colleghi, nel contestualizzare i dati salienti dell'attuale scenario macroeconomico, il DEF traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che il Governo intende attuare nel prossimo triennio. Si tratta del primo Documento che riporta in maniera organica e sistematica l'analitica descrizione delle linee programmatiche dell'azione dell'attuale Governo, al quale è affidato il non facile compito di riportare il nostro Paese su un sentiero di crescita economica, in un quadro di stabilità finanziaria. L'eredità pregressa non aiuta di certo a raggiungere l'obiettivo. L'economia italiana, caratterizzata dai bassi livelli di crescita registrati nel corso degli ultimi anni della pregressa esperienza di Governo, ha rivelato tutta la sua fragilità mostrandosi incapace, in un contesto economico internazionale ed europeo, che si è fatto progressivamente più difficile, di reggere ai contraccolpi di fattori esogeni quali il rallentamento dell'economia globale e il forte clima di incertezza nelle relazioni economiche internazionali. L'economia italiana ha registrato nel 2018 una crescita del PIL reale dello 0,9 rispetto all'1,7 per cento del 2017. A fronte di questi andamenti, nel quadro tendenziale, la previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 si attesta, secondo le ultime stime, attorno allo 0,1 per cento. Per quanto riguarda il PIL nominale, la stima tendenziale prevista per il 2019 si attesta all'1,2 per cento (0,2 per cento, se si tiene conto delle manovre messe in atto). Le prospettive di crescita dell'economia globale e del commercio internazionale, meno favorevoli, sono i principali responsabili della riduzione delle stime di crescita, soprattutto per quanto riguarda il 2019. In questo quadro, a prima vista negativo, manca ancora il contributo espansivo che le misure varate dal Governo nel corso dei primi dieci mesi di attività sapranno dare all'economia del Paese. Il Governo ha infatti realizzato alcune delle importanti misure contenute nel programma iniziale di riforma economica e sociale, come descritte nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, approvando il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di revisione del sistema pensionistico con quota 100. Attraverso l'erogazione dei benefici previsti dal reddito di cittadinanza sarà possibile imprimere un forte stimolo alla crescita dei consumi di beni primari. La misura assicura, infatti, un aiuto economico alle famiglie in difficoltà, che si distinguono per un'elevata propensione al consumo di beni di prima necessità. Questo comporterà l'immissione nell'economia reale di significative risorse destinate ad alimentare la crescita economica, grazie ad un elevato moltiplicatore del reddito, stante la bassa propensione al risparmio dei destinatari degli aiuti, senza contare i benefici legati all'attivazione di meccanismi virtuosi, quali i percorsi formativi e di accompagnamento all'inserimento lavorativo. Il Governo ha poi recentemente approvato due importanti misure contenute in altrettanti decreti-legge, che daranno un significativo contributo alla ripresa degli investimenti pubblici e privati e snelliranno le procedure previste per l'affidamento delle gare pubbliche. particolare attenzione: sono misure alle quali abbiamo fatto riferimento, ma che hanno un contenuto e una ripercussione di non poco conto. In particolare, il decreto crescita adotterà misure che favoriranno l'accumulazione di capitale e la realizzazione di investimenti produttivi attraverso misure come la reintroduzione del superammortamento, rimodulato per avvantaggiare le piccole e medie imprese, la riduzione delle aliquote delle imposte dirette applicate agli utili reimpiegati nel processo produttivo e la semplificazione delle procedure di fruizione di alcune agevolazioni. Il secondo provvedimento, il decreto-legge sblocca cantieri, citato nel DEF, punta a rinvigorire la ripresa nel settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti. Appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato e procedure di approvazione di varianti di progetto, l'aumento delle risorse destinate agli investimenti pubblici e agli incentivi per la ristrutturazione o ricostruzione degli immobili, anche in chiave antisismica, dovrebbero creare le condizioni per una vera ripresa di un settore che resta cruciale per l'occupazione e l'andamento generale dell'economia. Ma c'è un altro importante snodo della politica economica annunciata dal Governo con il DEF che mi rincuora ritrovare fra gli obiettivi prioritari dell'agenda di questo Governo della XVIII legislatura, per la prima volta, dopo l'avvicendarsi di numerose legislature. Mi riferisco al *welfare* familiare. Per troppo tempo abbiamo relegato a un ruolo del tutto marginale la famiglia e destinato ad essa interventi di natura assistenziale - quali il bonus bebè, ad esempio - con l'impiego di misure agevolative, fra loro disarticolate, che non hanno prodotto apprezzabili risultati in quanto prive di un approccio sistemico. L'Italia è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati e con una popolazione fra le più anziane. I dati contenuti nel rapporto annuale 2018 elaborato dall'Istat confermano che nel nostro Paese nascono ogni anno meno di 500.000 bambini e che il tasso di fecondità ha raggiunto il *record* negativo, che oscilla su valori di poco superiori all'1.34 figli per donna. Un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di due figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico. Il dato è di quelli che rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo futuro del Paese.

Avere un figlio è una risorsa in quanto incide positivamente sul PIL di 35.000 euro annui per ogni nuova nascita. Siamo di fronte a un inverno demografico; non possiamo chiudere gli occhi e far finta di nulla; il Governo sta manifestando la sua

I motivi che spingono i giovani a guardare con timore all'idea di procreare sono molteplici e gran parte di essi è legata alla sfera economica e alla mancanza di servizi e di efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme, non solo lavoratrici. Occorre superare la frammentazione degli attuali strumenti di sostegno, definendo politiche strutturali efficaci e incisive di promozione della natalità e dell'occupazione femminile, riordinando al contempo il sistema dei servizi e delle prestazioni sociali, anche al fine di definire un nuovo piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Inoltre, è fondamentale promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita familiare attraverso, ad esempio, ulteriori interventi sul sistema dei congedi di maternità e di paternità, favorendo favorendo la flessibilità del lavoro al fine di garantire alle famiglie la possibilità di provvedere in prima persona alla crescita dei propri figli; fattore - questo - che la comunità scientifica considera di estrema importanza per assicurare una crescita serena ai figli.

ormai da diversi anni, e confido nel fatto che tali propositi non vengano sacrificati sull'altare degli equilibri di finanza pubblica. Ne va del futuro dei nostri figli.

devo dire che ascolto con stupore crescente gli interventi di alcuni colleghi di maggioranza - tutti stimabili - ma ho la sensazione che il DEF non lo abbiano letto, perché altrimenti non credo potrebbero fare le affermazioni che fanno. politica ci ha abituati alla distanza che alcune volte c'è tra la propaganda e la realtà, ma con questo Governo non si parla di distanza: si parla di abissi, di iato iato enorme. Per mesi ci sono state parole, chiacchiere e propaganda; poi, a un certo punto, bisogna scrivere un documento: a farlo dev'essere un Ministro serio e competente,

lo stesso Governo ci dà ragione su tutto quello che abbiamo detto in questi mesi. Si tratta di una marcia indietro enorme, per l'assoluta consonanza tra i dati che troviamo nel DEF e quanto sostenuto da istituti nazionali e internazionali indipendenti, la verità è che i numeri alla base della legge di bilancio sono clamorosamente smentiti. Non so se provare tenerezza o rabbia per quella scena del balcone, in cui l'esultanza ridanciana del vice presidente Di Maio di fronte

anche se in cuor vostro sapete che sto dicendo la verità. Assistiamo a cose strane: sono al Governo e pensano di comportarsi come se fossero all'opposizione. Quando il ministro Tria ieri ha detto che, in mancanza di altre misure, sarà necessario aumentare l'IVA, una forza di opposizione avrebbe quando si sta al Governo, invece, bisogna dire «mai, perché invece faremo questo o quest'altro». *(Applausi dal Gruppo PD).* Quali sono le misure alternative che mettete in campo e le coperture? Siete al Governo: ditelo, se avete la possibilità di farlo. Il confronto tra le vostre previsioni programmatiche e il quadro tendenziale scritto nel DEF sarebbe esilarante, se non fosse drammatico: è tutto diverso da quanto prevedevate.

non si scherza sulla carne delle famiglie degli italiani (perché di questo si tratta, altro che battuta). Reddito di cittadinanza e quota 100 avrebbero dovuto determinare sorti magnifiche e l'aumento dell'occupazione: ora invece scrivete che il tasso di disoccupazione aumenterà dell'1,2 per cento, altro che tre posti di lavoro per ogni pensionamento; anche quella era una bugia. Veniamo ora, in conclusione, ad una materia maggiormente di pertinenza della mia Commissione, ossia gli investimenti in infrastrutture. Non è necessario essere uno scienziato dell'economia per sapere che, quando va male, bisogna investire in infrastrutture, grandi o piccole opere pubbliche e interventi classicamente anticiclici, evitando la chiusura di imprese, il fallimento dei grandi, dei piccoli, dei subappaltatori, dell'indotto e dei fornitori, nonché i licenziamenti. A fronte di tutto questo, invece,

dal quale non potevamo ovviamente esimerci. Quindi, fa piacere che ci sia un riconoscimento, da parte delle opposizioni, del fatto che questo DEF sia realistico e non ispirato a numeri inventati o alla propaganda,

che dobbiamo approvare pochi mesi dopo l'approvazione della legge di bilancio. È evidente che, a distanza di tre mesi, è impossibile avere un quadro effettivo dell'andamento dell'economia quest'anno è evidente che gli effetti della manovra non si sono ancora registrati nell'economia reale. È impossibile, ad esempio, che una delle scelte fondamentali di questo Governo, cioè l'investimento di forti risorse nel settore pubblico a favore degli enti locali

espressione e realizzazione completa nei tre mesi che sono trascorsi dall'approvazione di quei provvedimenti. È ovvio anche che la situazione è difficile, perché i dati dell'economia a livello internazionale e nell'eurozona in particolare sono preoccupanti e negativi. in cui questo Governo si trova ad affrontare la difficile partita del rilancio dell'economia è sicuramente peggiore e molto più grave di quello dei Governi precedenti. Però ci sono anche dei segnali positivi. C'è un dibattito su un dato rispetto alla produzione industriale: ci si chiede se il dato fornito nei giorni scorsi, relativo a una crescita della produzione industriale a gennaio e a febbraio, Io posso prendere in considerazione le obiezioni di tutti i parlamentari, come tutti noi possiamo fare, però il documento che ci è stato consegnato dall'ISTAT in audizione qualche giorno fa, proprio durante la discussione del DEF, testimonia un aumento della produzione industriale, che ad esempio a febbraio era dello 0,8 per cento, in controtendenza rispetto a tutti gli altri Paesi europei, Germania compresa. Questo dato ci è stato fornito ufficialmente e non credo che possa essere contestato in quest'Aula; è un piccolo segnale positivo, perché questo sì è un dato dell'economia reale e non è fondato su previsioni. È un dato che ovviamente ci fa ben sperare e che dimostra, al di là delle scelte economiche di questo o di quell'altro Governo, che c'è ancora un tessuto industriale molto forte e all'avanguardia nel nostro Paese; questo è sicuramente un dato positivo. poi un'altra scelta di questo Governo? L'abbiamo già detto: rimettere in moto l'economia attraverso la domanda interna. A fronte di una difficoltà a livello internazionale nelle esportazioni, l'immissione di denari a favore dei ceti medi e bassi della popolazione ha proprio questo scopo. Rispetto alle clausole di salvaguardia, ricordo che mai queste sono state disinnescate in un DEF e che mai si è detto con quale copertura sarebbero state disinnescate. ha l'impegno e il dovere di trovare il modo per disinnescare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA, e lo farà. Allo stesso modo ci siamo assunti l'impegno preso proprio dal ministro Tria in audizione - di trovare i 300 milioni per il trasporto pubblico locale. È un impegno che abbiamo preso e che manterremo. Sulla *flat tax* molto si è detto; è un obiettivo di questo Governo. Nella prima legge di bilancio è stata avviata una semplificazione e una riduzione fiscale per le partite IVA. A fronte del quadro economico, non la si poteva realizzare in un'unica soluzione, ma noi continueremo

invece, sosteneva che era impossibile superare la legge Fornero; ma noi l'abbiamo reso possibile. Qualcuno dichiarava di avere sfiducia rispetto alla nostra capacità di trovare risorse per gli enti locali; ma noi le abbiamo trovate. Quindi la strada è stretta, ma questo Governo ha la fiducia della maggioranza presente in Parlamento, alla Camera e al Senato. Ma la cosa ancora più importante è che ha la fiducia del Paese e della maggioranza dei cittadini, che noi quest'oggi confermiamo come Gruppo Lega,

sottoposto oggi all'esame di quest'Assemblea, ho subito pensato che sarebbe un atto di correttezza nei confronti del Parlamento e del Paese se, dopo la presentazione di questo DEF, qualcuno dai banchi del Governo avesse il coraggio di alzarsi e ammettere che ad ottobre, quando è stata presentata e approvata la nota di aggiornamento al DEF, hanno scherzato.

di aver fatto una battuta a suo tempo e che ovviamente in quel momento scherzava. Mentre a Palazzo Chigi c'è qualcuno che scherza e si diverte, il futuro del Paese oramai è ipotecato da una politica fatta di misure inconcludenti e di provvedimenti che, nel migliore dei casi,

Cari cittadini, è scritto nero su bianco nel DEF e non lo scrive l'opposizione, ma il Governo. Avremo crescita zero e *deficit* che sale. Lo ripeto: crescita zero e *deficit* che sale, certificato oggi

Famiglie e imprese oggi prevedono che a breve, soprattutto nel biennio 2020-2021, ci sarà un aumento della pressione fiscale dal 42 per cento al 42,7 per cento. Ciò avverrà - lo sapete benissimo perché è scritto nel DEF - per effetto dell'aumento dell'IVA e per effetto dell'aumento delle accise sulla benzina, che qualcuno aveva promesso

quindi di un Documento che possiamo definire assolutamente evanescente e fantascientifico, perché nel DEF non ci sono elementi essenziali per capire qual è il futuro del Paese e per comprendere quali sono gli obiettivi programmatici

ad aumentare il livello di occupazione dei giovani e delle donne. Invece il DEF certifica tutta l'inadeguatezza del Governo a gestire una fase e una congiuntura economica delicata e complessa, come quella che il Paese sta vivendo.

l'andamento previsto per le principali grandezze macroeconomiche, di cui forse non si è parlato abbastanza. Prendiamo il tasso di disoccupazione: si prevede che nel 2019 sarà più alto rispetto al 2018. La pressione fiscale: si prevede che nel 2019 sarà più alta rispetto al 2018. Il debito pubblico: si prevede che nel 2019 sarà più alto rispetto al 2018. *deficit* nominale: si prevede che nel 2019 sarà più alto rispetto al 2018. Il *deficit* strutturale: si prevede che nel 2019 sarà più alto rispetto al 2018. Allora viene da dire che questo, più che un DEF, ovvero un documento di economia e finanza, è un DFE, ovvero un documento di fallimento economico. C'è dell'irresponsabilità nelle forze che ci governano, perché si sta giocando con il futuro degli italiani. Non so come altro definire, se non un gioco irresponsabile, il teatrino il teatrino che è andato in scena e che temo continuerà ad andare in scena sull'aumento dell'IVA. Stiamo parlando di 23 miliardi di euro, che potrebbero scaricarsi addosso alle famiglie e alle imprese del nostro Paese. Stiamo parlando di un

catalogata come di secondaria importanza, ma non siete stati in grado di fare qualcosa di diverso dalle battute. Dire con voi l'IVA non aumenterà mai è una frase assolutamente priva di senso, se non si dice dove si troveranno i soldi per non farla aumentare. Sulle coperture non avete detto niente e tutti sappiamo che l'unica copertura che avete in mente, per non far aumentare

Qualcuno in Commissione ha detto che non si farà aumentare l'IVA tagliando le detrazioni fiscali, ma ciò significa non sapere di cosa si parla.

Quindi, il programma del Governo è evitare un massacro sociale, come l'aumento dell'IVA, facendo un altro. Capite che, comportandovi così, siete diventati produttori a getto continuo di incertezza, di sfiducia e di inaffidabilità. C'è qualcosa che dimostra che voi state facendo questo più di ogni altra, su cui forse non si è dibattuto abbastanza. Io vorrei fare ai rappresentanti del Governo, agli esponenti della maggioranza, al Ministro che è appena arrivato in Aula e che ci sta ascoltando questa domanda: nell'ultimo anno c'è un solo grande Paese europeo nel quale i tassi di interesse sui titoli pubblici decennali sono aumentati

Lo *spread* con la Germania, che tutti i giorni è all'attenzione delle cronache, ha l'andamento che sappiamo, ma non si dice dello *spread* con la Spagna, che ha un debito pubblico non molto diverso dal nostro, era 40 punti base un anno fa e 150 punti base oggi, e dello *spread* con il Portogallo, che era zero un anno fa ed è 140 punti base oggi. Questo avete fatto all'Italia e agli italiani e in questo DEF non notiamo alcun segno di ravvedimento. Fino a quattro mesi fa, ci avete fatto discutere - una discussione senza senso - di una stima di crescita per il 2019 di un punto e mezzo di PIL. Oggi ci venite a dire che il PIL crescerà dello 0,2, cioè avete completamente negato la stima che avevate fatto. Servirebbero delle riforme,

niente sul costo del lavoro, niente per la sburocratizzazione, niente per la velocizzazione della giustizia, niente di niente.

Si tratta di un passaggio importante, che ripercorre i risultati conseguiti in dieci mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio. Parliamo quindi di una cornice i cui contenuti saranno poi definiti in autunno, quando entrerà nel vivo la messa a punto della prossima manovra. Il DEF prevede nel programma di stabilità un *deficit* per il triennio 2019-2021 rispettivamente del 2,4, del 2,1 e dell'1,8 per cento in rapporto al PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, che è il vero valore di riferimento di cui si tiene conto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, il *deficit* strutturale è previsto nel triennio rispettivamente all'1,5, 1,4 e 1,1. Per il 2019, si avrebbe quindi un aumento del *deficit* strutturale di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione europea in relazione a spese straordinarie per il contrasto dei rischi idrogeologici ed interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello negativo dell' *output gap*, secondo il Governo il quadro programmatico per il 2019 assicura il rispetto del Patto di stabilità e crescita. Per gli anni successivi, il programma di stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il *deficit* strutturale fino a raggiungere lo 0,8 per cento del PIL nel 2022, in linea con la graduale convergenza verso gli obiettivi di bilancio concordati in sede europea. Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, esso è aumentato nel 2018 al 132,2 per cento e ne è previsto un aumento anche nel 2019, sino al 132,6 per cento. Il DEF ne prevede poi una riduzione a partire dal 2020, passando al 131,3

del patto di stabilità, sebbene prevedano miglioramenti più contenuti rispetto a quelli derivanti da un'interpretazione letterale delle regole del patto, come peraltro imposto dalle condizioni ancora difficili in cui versa l'economia italiana e il recente indebolimento ciclico. La ridotta crescita economica, infatti, non va addebitata al Governo, ma a un peggioramento del quadro economico globale, dovuto in particolare al conflitto protezionistico innescato dalla politica degli Stati Uniti, al rallentamento economico della Cina, all'instabilità provocata dalla Brexit e alla caduta della produzione industriale tedesca, alla quale la manifattura italiana è strettamente legata. Peraltro in Italia, in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei, negli ultimi mesi è stata registrata una crescita della produzione industriale che sta dimostrando la solidità del nostro settore manifatturiero. Nel dettaglio, i dati sulla produzione industriale italiana di gennaio e febbraio 2019 sono positivi, con una crescita rispettivamente dell'1,9 per cento e dello 0,8 per cento rispetto a dicembre 2018 e gennaio 2019. Passando al Programma nazionale di riforma, il Governo dimostra un'attenzione particolare all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione, con misure in favore del *welfare* familiare, della natalità e della genitorialità. Si prevede, inoltre, la valutazione dell'introduzione di un salario minimo orario, misura già presente in 22 Paesi su 28 dell'Unione europea. In più si continuerà a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione. In linea con il contratto di Governo, si intende inoltre continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi, la cosiddetta *flat tax*, e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel DEF. Il Governo prevede un rilancio della politica industriale dell'Italia, con l'obiettivo non solo di rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l'Italia protagonista in industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a standard ecologici più elevati rappresenta una vera opportunità di crescita per l'Italia, che deve essere perseguita attraverso l'incentivazione all'attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale nel nostro Paese. Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G, nella strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari. Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di accelerazione della crescita, che il Governo intende varare nei prossimi mesi e che procederà alla ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui. L'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. In questo contesto sono stati attuati interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, come la riforma organica delle procedure di insolvenza, cui si aggiungono le importanti risorse stanziate per risolvere le carenze di organico del personale amministrativo e della magistratura. Inoltre, l'Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità. Iniziative future verteranno, prioritariamente, sul riordino dei sussidi per la natalità, la genitorialità, la promozione del *welfare* familiare aziendale, il miglioramento del sistema sanitario e delle relative infrastrutture. Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell'azione di Governo, vi è anche il sostegno all'istruzione scolastica, universitaria e alla ricerca, attraverso misure atte

seriamente in considerazione le vostre proposte: il DEF di Tria, prudenziale, ma forse solo realistico, più che prudenziale; il DEF, invece, di fantasia, contenuto nella risoluzione dei due Vice *Premier*. Poi, facciamo anche una proposta. Perché noi le idee le abbiamo e le abbiamo anche piuttosto chiare. chiare. I dati vi sono stati detti più e più volte. Quello che stride moltissimo è che questo 0,2 per cento di crescita programmatica per il 2019 (dove crescita programmatica vuol dire la crescita che voi sperate di avere) fa molto sorridere, dal momento che quattro mesi fa irridevate i previsori nazionali e internazionali che prevedevano una crescita pari allo 0,6 per cento. Da questo punto di vista, dobbiamo tutti ammettere che la situazione è molto critica. Ovviamente tutto questo, avendo fatto una manovra espansiva del *deficit* ma non di crescita, incide sul *deficit*, incide sul rapporto *deficit*-PIL, incide sul rapporto debito-PIL.

saremmo nelle condizioni di dovercela cavare da soli, isolati politicamente e soli, senza strumenti di supporto da parte dell'Unione europea. europea. Tutto questo non può soddisfarvi. Noi, questa mattina, in Commissione finanze e tesoro siamo stati apostrofati come catastrofisti. Noi ci limitiamo ad essere realisti e ad essere preoccupati per il nostro Paese. Vorremmo tantissimo che lo foste anche voi. Vorremmo tantissimo che lo foste anche voi. Invece, non lo siete. Non lo siete, perché abbiamo sentito dire che questo collasso dei dati macroeconomici è dovuto al quadro internazionale. Certo, il quadro internazionale rallenta, l'eurozona rallenta, ma noi ci siamo fatti del male da soli. Abbiamo adottato delle misure inidonee a prevenire e a contrastare ciò che stava avanzando. Abbiamo fatto una politica di dichiarazioni di

Ma volete farne ancora perché la risoluzione di maggioranza che è un po' inconsistente, ne contiene degli altri. Vuole infondere questo ottimismo al Paese ma, in realtà, per chi la sa leggere, infonde

è stato detto, ironicamente, con una battuta da bar, che su 800 miliardi di spesa pubblica, 23 miliardi si trovano con facilità. Bene! Ma se fosse stato così facile, immagino che anche altri prima li avrebbero trovati. In ogni caso vogliamo sapere: dove? Vogliamo saperlo seriamente.

per cento del PIL. Noi abbiamo assoluto bisogno di crescita e di uno *shock*. Le donne sono lo *shock*, la risorsa preziosa che avete a disposizione del Paese. Usatela!

ma almeno di un ripensamento sull'impostazione della manovra 2019-2021, che voi avevate

Liberi e Uguali aveva presentato - vi avevamo pregato di affrontare un confronto con la Commissione europea per ottenere spazi, certo anche in *deficit*, ma per gli investimenti e per avviare - ad esempio - la transizione ecologica del nostro Paese. Questa mattina

ad insistere, pur nel clima di contrasto di questa lunga campagna elettorale, e vi apprestate ancora una volta a ripetere gli errori della manovra approvata l'anno scorso. In che senso? Spese correnti, *flat tax*, abbassamento ulteriore dell'aliquota IRES, pochissimi investimenti, tagli di spesa lineari, perché avete detto che non serve una manovra ma i 2 miliardi che avevate già previsto come clausola di salvaguardia che doveva entrare in vigore saranno applicati. Queste due linee

Ancora una volta, torno a ripetere, voi insistete su una politica fiscale iniqua, perché promettete vagamente la sterilizzazione degli aumenti programmati dell'IVA. Tutto questo è accompagnato anche da una miriade di riduzioni dei carichi fiscali e previdenziali, non sui lavoratori dipendenti ma sui lavoratori autonomi. Il quadro che ne esce è ancora una volta di

di effetti a soglia e anche una serie di piccole e varie *flat tax* che rischiano di far aumentare a dismisura anche l'elusione. Tutto questo a fronte anche della riduzione di gettito fiscale che queste misure, se adottate, implicherebbero. Parliamo poi della politica degli appalti.

in un quadro come quello realistico che avete fotografato, in un quadro di rischio di peggioramento a livello internazionale, noi non intravediamo assolutamente - e di questo c'era assoluta necessità un orientamento strategico, un asse su cui lavorare, una capacità di scelta, senza farsi troppo condizionare dall'esigenza a breve della ricerca del Ho citato prima la questione dei cambiamenti climatici. Noi continuiamo a dire che l'asse fondamentale consiste nell'avviare con forza e con determinazione la transizione energetica. Cercate risorse? Ma quando tagliate i 15-16 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi? Sono 16 miliardi che si possono recuperare e investire in un *green new deal*. Occorre insistere per la transizione energetica, per l'affrancamento dalla dipendenza dai fossili. Cercate tante risorse, ma questi continuate a confermarli e non si vede assolutamente una rinnovata capacità di fare un piano. A parole di piccole e grandi opere si discute tanto, ma in realtà su quel fronte la situazione degli investimenti rischia drasticamente di peggiorare. Noi non ci possiamo arrendere, perché prendiamo sul serio il fatto che non abbiamo più tempo,

che, magari passate le elezioni europee, potrà accadere qualcosa; ma non accade niente, se non si mette in campo una strategia diversa, con idee di responsabilità per la ripresa del cammino del Paese. La strada è quella disegnata: combattere i cambiamenti climatici. Salvare la vita umana sul pianeta significa avere la possibilità di salvare anche la nostra economia.

una politica economica produttiva. Dobbiamo a malincuore definire il DEF non come un libro dei sogni ‑ magari! ‑ ma come un manifesto elettorale, con

senza indicazioni precise sulle risorse. Cominciamo dal fantasma dell'IVA, dal giallo dell'IVA, su cui il Governo deve dire esattamente cosa vuole fare. Infatti, il ministro Tria

che le clausole di salvaguardia non si possono disinnescare perché non ci sono le risorse. È stato smentito da altre voci del suo stesso Governo, che hanno detto, fortemente e convintamente, che l'aumento dell'IVA non ci sarà.

che la risoluzione di maggioranza, con gli impegni di Governo, non risolve il giallo dell'IVA; essa, infatti, impegna il Governo, alla lettera *b)*, ad adottare misure per il disinnesco delle clausole fiscali di salvaguardia del 2020. comune buonsenso e senso comune, un po' di aria fritta, perché non contiene un'indicazione. Ma andiamo avanti. A nostro avviso, il Governo dovrebbe enunciare la propria politica economica e dovrebbe farlo in modo chiaro prima delle elezioni europee del 26 maggio, altrimenti ritorna il punto da cui sono partita, ossia che il DEF finisce per essere un manifesto elettorale. La verità, cari colleghi, è che questo Documento è frutto di misure assistenziali che pregiudicano intenzionalmente la competitività e i consumi. Il timore, anzi il rischio, è di vedere una stangata vera e propria abbattersi sulle imprese e sui consumi nel prossimo autunno. La certezza è che il Paese purtroppo è in recessione, che l'Italia ristagna. Il DEF sostanzialmente certifica la stagnazione. Il Governo, in nessuna riga di questo Documento, sostanzia

nel concreto, con una crescita dello 0,1 per cento del prodotto interno lordo, portando le previsioni del 2019, se tutto viene confermato, a un triste 0,2 cento, mi permetto di dire, con poca eleganza, con buona pace del decreto crescita e del neo bollinato decreto sblocca-cantieri. Fratelli d'Italia tiene a questa discussione perché ha una sua ricetta economica. Ieri la nostra *leader*, Giorgia Meloni, in un incontro organizzato dal collega Urso su impresa e lavoro ha ribadito davanti alle categorie produttive il nostro patto Noi abbiamo una ricetta, in parte contenuta nella risoluzione che abbiamo presentato, in parte nel programma elettorale delle europee e totalmente contenuta da sempre nel nostro DNA politico, che

più infrastrutture, più tutela del *made in Italy*, una riforma complessiva del sistema fiscale introducendo una vera *flat tax* per cento per famiglie e imprese sul reddito incrementale rispetto al periodo d'imposta precedente. Ancora, nella nostra ricetta proponiamo di destinare il 3 per

che queste considerazioni vanno contestualizzate con un ciclo internazionale economicamente critico, ma in Italia la pressione è più accentuata

Come non citare il reddito di cittadinanza che non risolve la povertà e non produce lavoro? E, ancora, la mancanza di investimenti pubblici, l'aumento della tassazione, la decrescita infelice per famiglie, aziende e per il sistema produttivo, con un quadro di debolezza economica italiana che incide evidentemente e negativamente sulla tenuta del sistema sociale, sulla coesione sociale. Non lo diciamo noi, ma lo dice l'OCSE, che ci ricorda che l'Italia rischia di chiudere l'anno in piena recessione con il calo del succitato 0,2 per cento nel economia europea con risultato così negativo. Sempre l'OCSE sottolinea, purtroppo, il fatto che l'Italia registra la minor crescita del PIL rispetto alla media europea. europea. In conclusione, ci sono economisti di fama internazionale che sulle fonti dell'OCSE, su queste constatazioni si chiedono addirittura - e lo sottolineo - se la scintilla della recessione globale arriverà dall'Italia ovvero se sarà l'Italia, insomma, a scatenare la prossima crisi globale. Quesiti importanti, enormi, di responsabilità. Io non so se sarà così, spero di no. Noi ci auguriamo che non sia così, perché siamo prima di tutto dei patrioti; amiamo l'Italia, amiamo questo Paese e ne vogliamo vedere la crescita felice. Tuttavia, devo dire quello che vediamo oggi non è un grande disegno economico, un Documento di programmazione economica. Quello che vediamo oggi è è un piccolo cabotaggio economico. Mi dispiace, ma questa non è la rotta di una navigazione che si utilizza per affrontare un pericolo superiore quale è quello che, purtroppo, si staglia di fronte all'Italia, di fronte a tutti noi.

Signor Presidente, colleghi senatori, Ministro, il bagno di umiltà, il ritorno con i piedi per terra del Governo - che questo DEF aveva lasciato intravedere in ragione di contenuti più prudenti - è durato poco. Troppo poco. Giusto un paio di giorni e poi ci siamo ritrovati travolti da un turbinio di dichiarazioni e di interpretazioni ardite, di versioni aggiornate del vergognoso microfono spento a lei, Ministro Tria: la volta scorsa era la Nadef, oggi il DEF. Il tutto per coprire - carta canta - quello che è stato già messo nero su bianco. Il vice ministro Castelli, ancora stamane in Commissione, ci ha detto testualmente che è un DEF scritto così, solo per sfuggire a una procedura di infrazione dell'Europa; come a volere ammettere di non poter dire la verità fino in fondo. Mi limiterò, allora, a fare due riflessioni. La prima riguarda la non coerenza dei quadri macroeconomici con i quadri di finanza pubblica.

salirebbe anche il tasso di disoccupazione all'11,1 nel 2020, e solo nel 2022, forse, tornerebbe ai livelli di inizio 2018: lo scrivete voi. voi. Come pensate di considerare questa ennesima stroncatura del decreto dignità? Tanto più che, per l'ennesima volta, siete proprio voi del Governo a scriverlo e a riconoscerlo. Non noi, ma voi. A fronte di questo, il *deficit* pubblico si dovrebbe portare quest'anno al 2,4 per cento del PIL, per scendere all'1,5 solo nel 2022. In sostanza, cancellate il miglioramento concordato con la Commissione europea per tornare al famoso *deficit* osannato dal celebre balcone. Ma, andiamo avanti. Il debito pubblico in rapporto al PIL aumenta al 132,6 per cento nel 2019 per poi scendere - nei quattro anni successivi - di uno 0,8 all'anno. Numeri che descrivono un quadro macroeconomico del tutto incoerente con quello di finanza pubblica. Delle due l'una: se aumenta l'IVA, così come è scritto nel DEF e come previsto dalle clausole di salvaguardia, così come confermato da lei, ministro Tria, in audizione - nonostante la contraerea di dichiarazioni immediatamente attivate immediatamente attivate - la crescita del 2020 andrà sotto lo zero (ovvero tra il meno 1 e il meno 2 per cento). Se, invece, non aumenta l'IVA nel 2020 - e ad oggi, come ha ben chiarito lei, Ministro, non ci sono misure alternative

PIL. Capite che così non reggiamo, vero, Ministro? Capite che questo è un quadro insostenibile per il nostro Paese? Paese? La seconda parte della mia riflessione riguarda gli effetti delle politiche economiche espresse direttamente dal Governo. Dal confronto tra gli andamenti tendenziali, che rispondono alla vostra prima legge di bilancio, e quelli programmatici, ovvero quelli che derivano dagli effetti che voi, Governo, attendete dalle vostre politiche economiche, sono pari a un impulso alla crescita dello 0,1 per cento

Non sorprende più, è vero, perché arrivate a fare anche di peggio. Questo minuscolo ed effimero impatto sulla crescita, che ha lo scopo di gonfiare ancora per un po' le vele del consenso, in realtà sgonfierà le tasche degli italiani, perché costa il peggioramento delle condizioni di *deficit* e debito pubblico: il primo è stato pressoché raddoppiato dalla vostra legge di bilancio e, di conseguenza, il debito crescerà di altri 150 miliardi di al 2022: dico 150 miliardi. Di fronte all'avanzare di un vero e proprio deserto economico, l'unico alibi che vi rimane è la scelta di aver presentato un DEF con un quadro di politiche invariate, lasciando l'aspetto programmatico ai provvedimenti da inserire nella prossima legge di bilancio, indicati ora nel DEF solo con generici titoli e senza alcuna quantificazione. se il buongiorno si vede dal mattino, sappiamo cosa ci aspetta: sono mesi infatti che vediamo licenziare decreti «salvo intese». Tornando ai vostri fiumi di parole, però, ci sono dati che indicano il netto peggioramento della crescita e dell'occupazione, il grave pericolo sul fronte dei conti pubblici e una prospettiva che a settembre richiederà una manovra di molte decine di miliardi di euro.

ma non può essere questa una giustificazione, perché tali analisi sono riferite esclusivamente al quadro interno e rispecchiano le vostre scelte di politica economica. Mi sia permesso qui, a conclusione, un breve accenno al Sud.

Dopo un quadriennio di sostanziale allineamento delle dinamiche economiche tra Nord e Sud, al Mezzogiorno tocca un peggioramento dello scenario di previsione, con una sensibile divergenza rispetto al Centro-Nord. La vostra tassa piatta, inoltre, è paradigmatica, perché avrebbe una ricaduta territoriale fortemente asimmetrica, a tutto svantaggio del Sud, l'area con i redditi più bassi. Stesso effetto avrebbe l'aumento dell'IVA: la scelta di lasciare il Mezzogiorno privo di politiche di sviluppo, quindi, è l'ennesima conferma dell'inutilità del vostro Ministero per il Sud, senza portafoglio né - cosa ben peggiore - uno straccio di progettualità per un bel pezzo d'Italia. Era e resta solo pura propaganda elettorale.

senza mascherarla con la demagogia e la propaganda e dicendo al Paese intero che siamo in piena stagnazione economica. La cosa più grave, signor Ministro, è che lei finalmente non solo dice *urbi et orbi* che i prossimi tre anni saranno saranno devastanti o molto critici per l'economia italiana, ma addirittura ci annuncia di dover incrementare l'IVA e le accise. Voglio dirle allora con estrema onestà intellettuale, signor Ministro, che non è un problema, perché i Governi che si sono succeduti prima di questo hanno inserito nei loro DEF l'eventualità di un incremento dell'IVA. Il problema sa qual è? È che fino a oggi nessuno all'interno solamente a lei) ci sta spiegando come vanno sterilizzate queste possibilità. Vede, questo alimenta il sospetto che purtroppo tramuta in una certezza l'eventualità di un incremento dell'IVA e delle accise. Fino ad oggi nessuno di voi ci ha spiegato come evitarlo; ci dite che lo eviterete, ci dite che dovremo passare sul vostro corpo, ma nessuno ci dice come farete. E lei finalmente oggi ci racconta la verità. Le dico un'altra cosa. Alcuni dei provvedimenti contenuti all'interno del DEF e che hanno raccontato il vostro primo anno ormai di Governo erano anche condivisibili o, quantomeno, il nostro approccio non è stato pregiudiziale. Penso al reddito di cittadinanza.

chiudete il sito «INPS per la famiglia», perché oggi è diventato ridicolo. Su tutti i giornali ci si sta chiedendo chi sono quei signori che rispondono in un modo quasi arlecchinesco a chi pone delle domande e si sente fuori

Quel reddito di cittadinanza - l'avevamo detto sin dall'inizio e lo abbiamo ribadito - non creerà alcuna occupazione (finalmente lo state costatando anche voi) e non inciderà sull'economia, tanto meno sui consumi, se non in una piccolissima percentuale. Vede, signor Ministro, non c'è nulla da fare. Mi rivolgo a lei, che è un economista e un accademico. Le regole per rilanciare l'economia sono le solite: più investimenti, meno lacci, più snellimento della burocrazia. Fino ad oggi - mi si permetta di dirglielo - non c'è nulla; c'è semplicemente la conferma di una visione statalista dell'economia italiana. E questo, come può vedere anche lei, non sta creando PIL, ma lo sta addirittura ponendo in una situazione drammatica. Gliel'ho detto ieri in Commissione e lo ribadisco oggi in Aula: noi non siamo delle Cassandre, ma riteniamo che, purtroppo per il Paese (perché l'instabilità non aiuta), questo sarà l'ultimo DEF di questo Governo. E questo - lo dico con molta sincerità - non per quello che è accaduto questa mattina, cioè per la vicenda che purtroppo colpisce un Sottosegretario della Repubblica. Mi rivolgo soprattutto agli amici della Lega. Vedete, per quanto il rapporto tra la Lega e i centristi negli ultimi tempi sia stato in nessuno di noi è mai balenata l'idea di archiviare e di non rimanere fedeli a quei principi di garanzia previsti dalla nostra Carta costituzionale. *(Applausi con i nostri alleati e con i nostri avversari. Siete voi, cari amici della Lega, che dovete porvi un quesito: è normale rimanere al Governo con chi da questa mattina, con uno stillicidio di dichiarazioni, non solo tende a denigrarvi, ma anche a delegittimarvi? Lo dico con molta franchezza agli amici del MoVimento 5 Stelle: qui non si tratta di essere più o meno garantisti, qui si tratta di essere omogenei nelle valutazioni. Quando c'è di mezzo qualche esponente dei 5 Stelle si adottano due pesi e due misure; la vicenda della sindaca Raggi oggi ce lo insegna. Vado a concludere, perché in sei minuti è difficile poter fare un ragionamento completo. Faccia però attenzione, signor Ministro: l'obiettivo di medio termine quest'anno è fissato a un + 0,5 per cento in più rispetto al pareggio di bilancio, mentre l'anno scorso era pari - 0,5 vuol dire che abbiamo l'1 per cento di PIL in più. Questo, senza entrare nel dettaglio, significa che i costi crescono per l'invecchiamento in questo Paese: più costa l'invecchiamento e la gestione dell'invecchiamento e meno risorse ci sono per le famiglie e per i giovani.

Ha presente? «Pane, amore e fantasia», la commedia di Vittorio De Sica. Gli italiani purtroppo dinanzi a loro avranno bisogno di tanta fantasia per poter contrastare le vostre scellerate politiche economiche.

Se vogliamo invece fare un'analisi, invece, più corretta e seria di quanto è successo e sta succedendo, dobbiamo partire innanzitutto dalle dichiarazioni del ministro Tria, che in audizione ha detto che, affinché l'Italia possa ridurre il *gap* di crescita con i *partner* europei, è anche necessario un cambiamento del modello di crescita europeo verso una promozione della domanda interna senza pregiudicare la competitività. Non dimentichiamoci che molte delle cause

non ha compreso minimamente che la stagnazione e la crisi del commercio mondiale erano dettate dalle politiche dei dazi americani, dalla Brexit - visto che ieri abbiamo votato il decreto - che non è stata capita fino in fondo e da tutte le conseguenze che ne derivavano perché sicuramente creava incertezza nei mercati, dall'aumento del prezzo del petrolio e dal rallentamento della Cina. Questi sono i fattori che stanno condizionando l'economia mondiale e non certo il Governo giallo-verde. Questo sia assolutamente chiaro. Bisognerebbe forse guardare le cose con un occhio più oggettivo, al di là della competizione e del confronto politico. Non si possono sempre usare questi toni, questi scenari apocalittici e queste previsioni catastrofiche della nostra economia perché, perché, alla fine, se andiamo a vedere i dati, non è proprio così tutto negativo come è stato dipinto. Vi ricordate i tanti interventi anche delle minoranze

La certificazione l'ha fatta Bankitalia perché, nonostante lo *spread*, le nuove emissioni sono a tassi inferiori rispetto ai titoli in scadenza. Insomma, la famosa spesa per interessi sul debito pubblico è calata di 1,7 miliardi tracollo del Paese, di politiche fallimentari del Governo e di conti pubblici alla deriva,

Vogliamo parlare della borsa? borsa? Anche la borsa ha la sua importanza. Citava bene oggi in Commissione finanze il collega Lannutti che ha detto che, da inizio 2019, la borsa italiana ha avuto i migliori risultati dell'Unione europea: in sei mesi ha fatto +13

Senatore Faraone, faccia il bravo. Gradirei sottolineare che anche sulla tassazione è stato detto in più di un'occasione

per come vi possono fare comodo. Dunque l'IVA non aumenterà. Se la sono presa con lei, ministro Tria, che però ha giustamente detto quello che sta scritto nel DEF, che è la fotografia del quadro attuale.

in un momento in cui c'è la crisi della domanda interna, ad aumentare l'IVA? Non aumenteremo l'IVA, ma quello che è certo, visto che si parla dell'IVA, è che se c'è stato un Governo che l'ha aumentata è il Governo Letta nel 2013.

Adesso proseguiamo, non per i ricchi, ma per il ceto medio, fino a 50.000 euro di reddito familiare. Questa è l'impostazione iniziale e indubbiamente non andiamo a favore dei ricchi, ma

che vanno semplificati, anche e soprattutto per una ragione. Perché erogare questi sconti e questi *bonus* - ho letto e ha detto bene il vice ministro Garavaglia - costa anche un sacco di soldi allo Stato. Forse è allora meglio ridurre le tasse, recuperare delle risorse e finalmente aiutare le nostre famiglie, che è quello che vogliamo tutti noi.

vi stupiremo anche nei prossimi trimestri.

colleghe e colleghi, il Governo ci sottopone un Documento di economia e finanza per il 2019 prudenziale, visto il momento congiunturale di rallentamento economico a livello globale e il minore dinamismo del commercio internazionale. La crescita è stata rivista al ribasso dalle principali economie mondiali e, per fare un esempio, la Germania sta passando da una previsione di crescita dell'1,9 per cento a una dello 0,5 per cento: una riduzione nettamente superiore alla nostra. Questo DEF prevede una crescita dello 0,2 per cento per il 2019, frutto anche di un aumento della spesa per investimenti e dell'effetto del reddito di cittadinanza. Per l'anno successivo si prevede un incremento del PIL dello 0,8 per cento. Troppo poco? Potremmo anche dare una risposta affermativa, ma dovremmo farlo, come detto, con l'obbligo di tenere in considerazione un contesto di difficoltà generale. Piuttosto, ci sono alcuni elementi che ci inducono a ben sperare: il potere d'acquisto delle famiglie aumenta dello 0,9 per cento rispetto al 2018; aumenta finalmente, dopo anni di calo, la propensione al risparmio; riprendono ad aumentare i consumi dopo una sostanziale stagnazione negli ultimi due trimestri del 2018; aumentano anche la produzione industriale nel primo bimestre dell'anno, come certificato da Istat e Bankitalia, e la fiducia delle imprese. Di tutti questi dati macroeconomici hanno già parlato diffusamente le colleghe e colleghi che mi hanno preceduta. Quello su cui vorrei soffermarmi, dunque, è l'impatto sulla vita reale di tutti questi numeri. Ebbene, allegati al Documento di economia e finanza ci sono gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), una serie di indicatori che ci dicono se e come migliora la vita dei cittadini italiani in base alle politiche messe in atto dal Governo. In pratica, il riferimento è a cosa toccheranno effettivamente con mano gli italiani, aspetto che dovrebbe costituire il primo pensiero della classe politica e che di sicuro è il nostro. La prima cosa che influenza positivamente gli indicatori di BES è la forte concentrazione di risorse finanziarie sui numerosi aspetti che attengono all'inclusione sociale. È stata infatti finalmente prevista l'adozione di misure volte a contrastare la povertà, incrementare il reddito disponibile delle famiglie, favorire la partecipazione al mercato del lavoro, la formazione e il ricambio generazionale, stimolare gli investimenti (anche per l'efficienza energetica), fornire agevolazioni fiscali al tessuto produttivo ed in particolare a professionisti e piccole imprese, sostenere la ricerca e rafforzare la sicurezza dei cittadini. Ed infatti aumenta il reddito medio disponibile e si riducono l'indice di disuguaglianza e quello di povertà assoluta. Tutto sostanzialmente grazie all'introduzione del reddito di cittadinanza. Per questo trovo inconcepibili i continui e ripetuti attacchi rivolti a questa misura, addirittura definita da una sigla sindacale durante le audizioni una ricetta sbagliata che va cambiata. come si fa a parlare di misura sbagliata se è appena entrata in vigore e le prime risposte stanno arrivando ai cittadini in questi giorni? A mio avviso è solo pregiudizio e opposizione senza motivo *(Applausi dal senatore Saviane)*, se non quello della perdita di controllo che si vorrebbe continuare ad avere sulle fasce deboli della popolazione, che invece in questo modo possono affrancarsi È evidente come il Governo sia al lavoro per migliorare l'inclusione sociale, contrastare il precariato e incentivare il lavoro giovanile e femminile grazie alle misure in materia pensionistica e al reddito di cittadinanza, interventi che verranno completati dall'introduzione del salario minimo orario. Un collega che mi ha preceduto ha detto che presto gli italiani si accorgeranno dell'errore fatto nel votarci. Gli rispondo che per adesso circa 500.000 famiglie si stanno accorgendo che il reddito di cittadinanza è realtà, perché stanno già arrivando a casa le *card* con gli importi spettanti caricati e che potranno quindi immediatamente essere spesi. M5S)*. Dicevo che grazie alle politiche del nostro Governo migliora il rapporto tra tasso di occupazione delle donne tra venticinque e quarantanove anni con figli in età prescolare e delle donne di pari età senza figli; migliora poi l'efficacia della giustizia civile; si riducono, invece, la criminalità predatoria e l'abusivismo edilizio. Anche in campo ambientale stanno per essere varate norme importanti che porteranno ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica: misure per incentivare la produzione energetica da fonti rinnovabili (i decreti ministeriali ministeriali FER 1 e FER 2); l'attuazione del piano strategico della mobilità sostenibile, che prevede il rinnovo del parco bus, il rafforzamento del trasporto pubblico, l'incentivazione della riconversione del parco delle auto private con mezzi a basso impatto emissivo. Certamente ci sono campi dove dobbiamo fare ancora di più, come l'ambito sanitario e l'istruzione, ma il Programma nazionale di riforma identifica le principali misure da intraprendere in aggiunta a quelle già previste nella legge di bilancio 2019. conclusione, ritengo positivo il quadro delineato dal Governo in questo Documento di economia e finanza in discussione; penso che il clima di fiducia che già si inizia a respirare non potrà che migliorare man mano che si inizieranno a vedere gli effetti delle misure varate e saranno approvati gli altri provvedimenti previsti. Aggiungo che è un dato che dimostra la maggiore fiducia anche l'aumento della disoccupazione, perché aumenta per effetto del passaggio degli inattivi a disoccupati, ossia a persone in cerca di occupazione; persone che dallo scoramento totale tornano ad avere una speranza nel futuro e a cercare lavoro;

a milioni di italiani grazie alla presenza del MoVimento 5 Stelle alla guida del Paese. Dichiaro aperta la discussione

La Presidenza prende atto che i relatori di maggioranza e di minoranza hanno rinunciato alle repliche in ragione dei tempi stretti

Patuanelli e Romeo. Decorre pertanto da questo momento il termine di trenta minuti per presentare eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Signor Presidente, cercherò di essere breve, anche perché molte questioni sono state già discusse, e cercherò di evitare di dare i dati, che sono stati citati più volte. Consentitemi, però, qualche commento anche a questi dati. Questa discussione è importante, perché il DEF 2019 riporta i risultati conseguiti in questi dieci mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio. Richiamo il contesto economico, che è stato più volte qui richiamato e dibattuto. delle correzioni progressive delle previsioni economiche fatte dal Governo, fino ad arrivare alla previsione dello 0,1 per il 2019, come previsione tendenziale, e dello 0,2, come obiettivo programmatico,

apportate al tasso di crescita, anche della Germania, siano state ancora più forti. È stato quindi richiamato - o forse

restringimento del *gap* di crescita dell'Italia rispetto all'eurozona molto forte.

si ridurrà allo 0,6 rispetto alla eurozona e, addirittura, allo 0,5, rispetto alla Germania. Ma, nello stesso tempo, peggiorano le previsioni previsioni di crescita per la Germania. Ovviamente, non era questo restringimento del *gap* di crescita che noi cercavamo, quando abbiamo posto l'obiettivo un anno fa. Vi ricordo, infatti,

Evidentemente, ci troviamo in una situazione complessa per l'economia italiana, per l'economia europea e anche per l'economia a livello globale. è responsabilità del Governo questo rallentamento, ma certamente è responsabilità del Governo la reazione a questo rallentamento del tasso di crescita. allora porci la domanda: quale dovrebbe essere la reazione? Dobbiamo cambiare la strategia, dopo appena tre mesi dall'approvazione della legge di bilancio? Se le circostanze lo richiedono, bisogna avere il coraggio di cambiare strategia. Ma quali erano i pilastri della strategia che noi abbiamo posto all'azione di Governo? Investimenti pubblici a supporto anche degli investimenti privati; aumentare il rendimento del capitale in Italia per questa strada; portare un ammodernamento di tutte le infrastrutture tecnologiche e di trasporto, anche di quelle immateriali e, in questo modo, aumentare la competitività dell'Italia. Questo era l'obiettivo. L'opposizione dirà - come ha detto

accumulati negli anni in una struttura regolatoria complessa, consentita dai Governi che ci hanno preceduto e anche dal decadimento della capacità tecnica della pubblica amministrazione. Il secondo punto era rappresentato dalla riforma fiscale e dall'attuazione progressiva di un sistema di *flat tax*, che è iniziato quest'anno.

anche perché - forse è stato richiamato - è necessario discutere, in questa complicata fase dell'economia italiana ed europea, del cambiamento del modello di crescita, di cui si discute oggi anche a livello europeo. Voglio dire che i tre punti richiamati - rilancio degli investimenti pubblici; riforme fiscali; rafforzamento delle reti di protezione sociale e provvedimenti di inclusione sociale - sono al centro del dibattito internazionale ed europeo, perché la situazione è cambiata. I fatti dell'economia stanno conducendo a un dibattito anche in Europa e a livello internazionale su tali questioni. In ottobre era difficile parlare di questo, il mondo si concentrava nella discussione su quali potevano essere

fase ci dice che nella prima metà dell'anno avremo un tasso di crescita molto basso, ma i primi dati dicono che siamo in territorio positivo. Poco fa la Banca d'Italia ha detto che si riprende

Per gli anni successivi vi ho citato le previsioni non solo nostre, ma anche del Fondo monetario internazionale. In questi mesi l'opposizione non ha fatto altro che dire che, di fronte alla difficoltà dell'economia, era necessaria una manovra correttiva. Ho sempre detto che non si sarebbe fatta alcuna manovra correttiva. *(Applausi dai Non l'abbiamo fatta perché era evidente che, di fronte a un rallentamento forte dell'economia, non si fanno manovre fiscali restrittive. Questo non lo chiedeva neppure l'Europa; lo si chiedeva solo qui. Ovviamente, poiché, come si dice in gergo, non abbiamo molto spazio fiscale e bisogna mantenere

il rapporto tra debito e PIL. Voglio richiamare che l'obiettivo di discesa del rapporto debito-PIL nel DEF reso in modo chiaro per il prossimo triennio. Al tempo stesso, voglio anche dire che il nostro debito - e noi dobbiamo dirlo, credo, tutti uniti al mondo - è perfettamente sostenibile. *(Applausi In una fase di caduta del tasso di crescita, non siamo di fronte all'esplosione del debito. Negli ultimi anni il nostro debito si è stabilizzato: qualche anno cresce un pochino, qualche anno diminuisce un pochino. Ovviamente, il problema è metterlo su un sentiero di decrescita costante. In questa fase è complicato ovviamente, ma è questo l'obiettivo per il prossimo triennio. Per questo, nel prossimo triennio abbiamo fissato degli obiettivi chiari

Non solo non c'è manovra correttiva, ma abbiamo fatto un po' di manovra correttiva in senso contrario, perché i due decreti che stanno per essere varati portano portano poche risorse aggiuntive, ma importanti, perché ben indirizzate al sostegno degli investimenti. Poche risorse aggiuntive perché dobbiamo mantenere gli obiettivi di finanza pubblica (abbiamo utilizzato, in parte soltanto, alcuni risparmi che avremo anche sul pagamento degli interessi) ma tutti i provvedimenti vanno nella direzione di un sostegno alle imprese, al credito, alle piccole imprese, a sostenere gli investimenti in un momento in cui sono difficili, per via della congiuntura internazionale: quando non ci sono ordinativi, è difficile che le imprese facciano investimenti. ci sono seri provvedimenti per iniziare a smontare quell'impalcatura che nel codice degli appalti blocca, in molta parte, la rapidità con cui i fondi di investimento pubblici diventano effettivamente effettivamente cantieri. Quindi è una manovra correttiva in senso contrario, perché stiamo reagendo. L'impatto ovviamente per cento, perché partiamo a metà anno, ma può essere significativo anche negli anni successivi. Tutte le previsioni sono abbastanza prudenti. Voglio richiamare anche il fatto che, quando si parla di aumento del tasso di disoccupazione, bisogna bisogna leggere anche l'ultima riga della tabella sul tasso di disoccupazione; è chiaro che c'è un effetto statistico anche iniziale, perché, con il reddito di cittadinanza, prima fase ci saranno centinaia di migliaia di persone che entreranno nella forza lavoro, e statisticamente questo significa aumentare immediatamente il tasso di disoccupazione, prima che poi questo si traduca in un

il numero degli occupati si riduce e c'è un tempo per sostituirli; qualunque sia il tasso di sostituzione previsto, in ogni caso ci vuole un certo tempo, quindi abbiamo questo effetto immediato. Ma diamo conto anche di questi dati. Questa è la situazione. C'è una strategia? Sì. C'è una strategia che riguarda la conferma delle manovre che sono state approvate con la legge di bilancio 2019, delle manovre aggiuntive, e poi ci sono questi obiettivi di finanza pubblica. E qui vengo al punto su cui si discute ogni giorno: l'IVA. Questo DEF in gran parte, sostanzialmente, accetta il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. E a legislazione vigente, come è scritto nel DEF, c'è l'aumento dell'IVA, che non è una clausola di salvaguardia, perché le clausole di salvaguardia sono proibite dalle leggi di contabilità. È una legge, che dovrà essere cambiata per evitare, se vogliamo prendere una decisione politica, l'aumento dell'IVA. Questo problema verrà affrontato quando si disegnerà la legge di bilancio del 2020, assieme alla continuazione di un altro *step*, di un altro passo, della riforma fiscale presente nel programma di Governo. Ciò significa che bisogna trovare le risorse per farlo; ma questa è una tautologia, evidentemente, nel momento che in questo DEF si fissano gli obiettivi di finanza pubblica e nel DEF che la manovra che si farà con la legge di bilancio nella direzione di evitare l'aumento dell'IVA e di continuare nella riforma fiscale, muovendo un altro passo in quella direzione, verrà fatta nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo DEF. D'altra parte, nella seconda metà dell'anno noi avremo molte altre informazioni. In primo luogo, l'informazione su quale sarà l'evoluzione effettiva dell'economia italiana, che ‑ ripeto ‑ dipende molto da come reagiranno la Germania e le altre parti dell'Europa al rallentamento, perché potremmo avere uno scenario più negativo o uno più positivo. L'unica previsione che si può fare ‑ l'ho già detto ‑ con cui sempre si indovina è che le previsioni poi cambiano; cambiano; dobbiamo quindi vedere quale sarà la situazione macroeconomica e disegnare, in funzione della crescita economica, quello che faremo. Avremo anche i dati, quelli sì, inizialmente effettivi, sull'andamento della spesa per le misure che abbiamo adottato con la legge di bilancio per il 2019, in primo luogo il reddito di cittadinanza e quota 100. Stiamo monitorando e monitoreremo la spesa e in autunno avremo una valutazione più chiara di quali saranno gli andamenti. Vedremo anche se saremo riusciti a far ripartire

cui penso sia importante, poiché il momento è difficile, che tutti guardiamo alle questioni di fondo: se si faranno queste cose, se riusciremo a far ripartire gli investimenti pubblici, se i provvedimenti che stiamo adottando in questi giorni riusciranno veramente a sbloccare i cantieri. Queste sono le questioni di fondo per agire. È chiaro, poi, che l'economia, compreso il settore privato, deve reagire e non seguire soltanto un modello, quello tedesco, che sta entrando in crisi. Da questo punto di vista, anche il rilancio della domanda interna è un problema di tutta l'Europa.

Signor Presidente, signor Ministro, esprimo la mia posizione favorevole sul DEF presentato dal ministro Tria e validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale peraltro ha correttamente evidenziato rilevanti rischi di crescita inferiore a quella prevista, già molto modesta. Rispetto alle proposte di risoluzione presentate, mi riservo di orientare il mio voto dopo averle attentamente lette. Se mi pronuncio favorevolmente è perché interpreto questo DEF non tanto come Documento di economia e finanza, con una visione credibile e una strategia concreta per ridare dinamismo all'economia e alla società italiane, cose che, malgrado gli sforzi, non vedo, ma perché quest'anno, a mio giudizio, l'acronimo DEF va inteso in un altro modo: dichiarazione di evitato fallimento. Non lo dico in senso denigratorio, al contrario. Infatti i cittadini italiani devono essere grati al ministro Tria, mite ma coriaceo, capace di resistere a dosi illimitate di derisione, di assorbirle con espressione sorridente, di porgere sempre l'altra guancia. A volte mi sono chiesto con un po' di stizza: «Ma quante guance ha quel Ministro?». Il Ministro dell'economia e delle finanze è riuscito ad attenuare gli effetti, per certi aspetti potenzialmente fallimentari per la finanza pubblica, oltre che negativi per la crescita, che la politica economica del Governo a briglie sciolte avrebbe provocato. Allo stesso modo, guardando avanti, questo DEF a profilo basso ha almeno un pregio: ricorda ai cittadini - e osa perfino ricordare ai governanti - che tutto non si può contemporaneamente fare. L'aumento dell'IVA certo sarebbe regressivo e recessivo, secondo come inopportunità solo al taglio delle agevolazioni alle fasce più deboli della società: cito questo perché fu il dilemma di fronte al quale mi trovai a fine 2011, quando ereditai dal Governo precedente la prima clausola di salvaguardia, introdotta in situazione già di emergenza finanziaria nell'agosto del 2011, per 20 miliardi. Riuscimmo a disinnescarla per 13,4 miliardi, ma il resto andò in un punto di aumento dell'IVA, a malincuore e solo perché sarebbe stato ancora peggio, credo, economicamente e socialmente, tagliare le agevolazioni alle fasce socialmente più deboli. In questa fase politica e di dibattito pubblico che attraversiamo credo che sia grande merito del Ministro mettere in luce che tutto non si può fare, che ogni cosa ha i suoi costi e che le risorse sono limitate. sono convinto che lo sia dai cittadini ma, se mi posso permettere, i membri dei partiti della maggioranza e il Governo, secondo me, dovrebbero rispettare ancora di più un Ministro che, in modo serafico e presentandola come tautologia, riesce a rappresentare il fatto che le risorse sono limitate e che dei vincoli di bilancio esisterebbero persino senza l'Unione europea, solo per il fatto che abbiamo dei figli, dei nipoti e che ci sono le generazioni future. la mia posizione su questo DEF un po' sommesso è favorevole, soprattutto perché può servire come chiarimento a chi governa e all'opinione pubblica, che deve seguire le mosse di chi governa e delle opposizioni, che hanno avuto tanti validi argomenti oggi, per muoversi in una concretezza di scelte limitate dalle risorse.

a soli sei mesi dalla Nota di aggiornamento in cui si parlava di una crescita per il 2019 dell'1,5 per cento, oggi il Governo certifica che questa è appena dello 0,2. Inoltre, nelle previsioni di questo DEF si evidenzia come le misure bandiera del reddito di cittadinanza e di quota 100 non porteranno alcun miglioramento all'andamento attuale dell'economia. Questo vuol dire due cose: che l'Italia è sull'orlo della recessione economica e che questa recessione è il risultato anche di politiche profondamente sbagliate. Eppure, il rallentamento del quadro internazionale indicava la strada già dallo scorso anno: tutelare l'andamento positivo degli ultimi trimestri mettendo le risorse a favore delle imprese e del sistema produttivo, abbassando la pressione fiscale per il ceto medio. Come tanti altri abbiamo subito espresso la nostra perplessità per le misure bandiera. Adesso è chiaro a tutti: o bisognerà tagliare i servizi pubblici o aumenterà l'IVA per finanziarli.

subiranno un duro colpo sulla competitività. L'IVA ordinaria in Austria é al 20 per cento, 5 punti in meno di quella che ci sarà in Italia con l'eventuale aumento. Come se non bastasse, il Governo annuncia di voler introdurre la *flat tax*, una misura tutta a vantaggio dei ceti abbienti. Non si capisce come si possa prospettare la *flat tax* in questo quadro così difficile; non c'è la minima possibilità di finanziarla. Di certo, non sarà sufficiente la cancellazione degli sgravi e delle deduzioni fiscali, che comunque sono strumenti importanti perché servono a indirizzare la società a comportamenti desiderati. In conclusione, aumentare l'IVA e introdurre la *flat tax* è in netto contrasto con la narrazione portata avanti in questi mesi di un Governo attento agli ultimi e interessato a rilanciare i consumi con quota 100 e il reddito di cittadinanza. Spero davvero che, una volta superato il 26 maggio, sapremo qualcosa di più sulla programmazione. Ad oggi non è chiaro a chi verranno tagliati i 2 miliardi di clausola in uscita. Non si sa che fine abbia fatto il piano di privatizzazioni con cui il Governo contava di recuperare

Il punto vero è che, ancora una volta, questo Governo si dimostra del tutto irresponsabile e guidato solo da obiettivi di carattere elettorale. Comprare consensi aumentando il debito pubblico vuol dire governare il presente scaricando i costi sulle future generazioni. Si tratta del più grave dei problemi, proprio come ha spiegato la giovane Greta oggi, qui in Senato. Per questo motivo, il nostro Gruppo voterà contro la risoluzione presentata dalla maggioranza.

forse aveva ragione il presidente Conte quando ci ha detto che i tempi di questo DEF, in un quadro di così grande incertezza, non sono proprio quelli più adeguati. Sì, perché il quadro, oggettivamente, è molto serio e molto critico. Tuttavia, da qui a un documento - ministro, Tria - che non dà alcuna risposta e senza alcuna indicazione, ci sta tutto l'imbarazzo del Governo. A questo punto, non solo viene da pensare che si è deciso di rinviare ogni scelta a dopo le elezioni, per poter raccontare così tutto e il contrario di tutto già questo sarebbe molto grave - ma forse il problema è la mancanza di una strategia: non c'è un disegno per il Paese, solo *spot*,

In verità, l'unica cosa che tiene insieme 5 Stelle e Lega non è il contratto; io temo che sia la gestione del potere. Lo stiamo ravvisando in modo clamoroso: non siamo di fronte a una rivoluzione, siamo di fronte a una rivoluzione mancata, a promesse e racconti lontanissimi dalla verità. Il quadro dei numeri è realistico: Ministro, non potevate fare diversamente, diciamoci la verità. Non potevate scrivere altri numeri, vista la valutazione. Ci avevate già provato nella legge di bilancio

o no? Ancora, sarei prudente: anch'io vorrei, come voi, che la ripresa della produzione industriale in questi due mesi si consolidasse e crescesse,

anzi, affrontare la questione della legge Fornero era ed è essenziale, ma il problema è che voi non l'avete abolita, avete fatto semplicemente un nuovo scalone. Non penso che le persone vogliano stare sul divano: vogliono lavorare, ma voi continuate a confondere il lavoro con interventi sulla povertà. Ci sono poi i decreti-legge crescita e sblocca cantieri,

per le questioni di legalità che si apriranno, se le notizie sono corrette. Il problema vero è che, come vi ha detto giustamente il Presidente della Repubblica, non si può tenere

Ora, invece di scrivere quello che avete affermato nella risoluzione, scrivete chiaramente: «L'Iva non aumenterà», perché non l'avete fatto nella vostra risoluzione.

Come si affronteranno questi problemi? Non chiedo una tabella, non la chiedevo nel DEF. Come si affronteranno questi problemi non ce lo avete detto e non è che non lo avete detto solo al Senato o alla Camera, non lo dite agli italiani, non lo dite agli italiani, che avrebbero piacere di saperlo perché si tratta di un problema che riguarda le risorse che, per usare una vecchia espressione,

dire, e gli annunci che avete fatto non stanno in piedi. Ora, io vorrei dire in modo molto chiaro siamo isolati dall'Europa. Sono d'accordo che deve cambiare la politica europea, ma non ce la farete mai se continuerete a sbattere i pugni sul tavolo e a insultare mezza Europa: non cambierà mai l'Europa; non cambierà mai.

della spesa, non c'è un principio. Le tre voci più importanti sono: pubblica amministrazione, sanità e istruzione. Vediamo come siamo messi. Qui c'è un grandissimo problema, nella pubblica amministrazione c'è un'emergenza: mancano insegnanti e medici. La Corte dei conti dice che nel vostro DEF manca nel vostro DEF manca la copertura dei contratti, figuriamoci quelle migliaia e migliaia di assunzioni che bisognerebbe fare. proponete investimenti. Ora, guardiamo un attimo questi investimenti: avete

ma se non assumiamo nei Comuni, nelle Regioni e nelle Province personale specializzato per fare gli appalti, tutto rimarrà bloccato.

Non parlate e non si affronta una questione drammatica come quella del Mezzogiorno e magari volete fare l'autonomia differenziata senza principi fondamentali: il federalismo «fai da te» darà un colpo all'intero Paese e, in primo luogo, al Mezzogiorno. Avete un problema serio (fatemi concludere così): invece di fare cabine di regia e strumenti centralizzati che non funzioneranno, un grande problema di coordinamento ce l'avete. Il Presidente del Consiglio ce l'ha: deve spiegare al Ministro dell'interno che non può essere Ministro dell'interno, Ministro dell'economia, Ministro della difesa, Ministro degli affari esteri e non può essere il sindaco di tutti i Comuni italiani. È un problema di Costituzione.

che il già presidente del Consiglio Monti ha dato un giudizio positivo di questo Documento di economia e finanza. Il già presidente del Consiglio Monti ha detto che questa è la strada giusta, prefigurando quello che è nelle sue cognizioni politiche e finanziarie e che gli italiani già ben conoscono. Lo dico non soltanto agli amici della Lega e ai colleghi dei 5 Stelle, lo dico agli italiani: cosa è successo in questi dieci mesi, se il presidente Monti, colui che ha realizzato manovre economiche che purtroppo hanno penalizzato l'Italia produttiva e l'Italia sociale, è giunto a un giudizio positivo di questo Documento e delle prospettive che realizza? lo chiamo "*premier*"), che un anno fa, prima di fare il Governo, prospettava per l'Italia una manovra economica che quest'anno avrebbe portato a un +2,5 Lo dico alla maggioranza, che pensava di realizzare una manovra economica pari all'1,5 e che poi, ancora quattro mesi fa, parlava di una crescita dell'1 per cento. Lo dico al presidente del Consiglio Conte, che parlava di un anno bellissimo e chiedo agli italiani che ci stanno ascoltando se questo è il loro anno bellissimo. Lo dico al vice *premier* Di Maio, che ha le leve economiche del Paese e che ancora l'11 gennaio di quest'anno parlava del nuovo miracolo economico italiano che in primavera si sarebbe sviluppato e chiedo ai cittadini italiani se siamo di fronte a un nuovo miracolo economico italiano. Cos'è accaduto? È accaduto che avete fatto una manovra economica del cambiamento additando a tutti che il nemico erano l'Europa e le sue regole e oggi vi adattate pienamente alle regole europee. Avete detto che avreste sforato le regole europee e poi avete contrattato pietosamente, già nella manovra economica di bilancio, un mero +1 per cento. Ministro Tria, accanto a lei non c'è il Ministro per le politiche europee. Perché non c'è? Dov'è finito il ministro Paolo Savona, che avrebbe dovuto cambiare con voi l'Europa? Si è dimesso dal Governo e non l'avete sostituito: non abbiamo nemmeno chi ci rappresenta nell'Unione europea! Vi siete arresi. Avete dipinto allora che il nemico era l'Europa e quest'anno ho sentito i discorsi dei colleghi della maggioranza, che dicono che ora non c'è solo l'Europa contro l'Italia, c'è anche la Germania che si è arrestata, c'è anche la Cina che cresce meno, ci sono anche gli Stati Uniti e c'è persino il Regno Unito con la Brexit, ci sono il Brasile e l'America latina che non crescono: il mondo è contro di voi. Il prossimo anno a chi Il prossimo anno a chi darete la colpa della recessione, della disoccupazione, del calo dei consumi, del calo degli investimenti e dell'aumento della povertà in questo Paese? La darete ai marziani la colpa? O vi assumerete le responsabilità di ciò che avete determinato con una manovra economica fallimentare a cui, come ha detto oggi il ministro Tria,

Non c'è nulla nel Documento di economia e finanza, ancorché vi siano spese complessive per circa 133 miliardi di euro nei prossimi tre anni anni e, soltanto per quest'anno, 23 miliardi di euro da recuperare per evitare l'aumento dell'IVA e 400 milioni di euro per evitare l'aumento delle accise sulla benzina, che avevate detto che avreste cancellato.

se aumenterete l'IVA, come vi ha suggerito Monti, comunque, perché lui questo ha fatto, se metterete una patrimoniale, di cui parlate nelle vostre congreghe riservate. Non dite più nulla; non avete più un sogno, non avete un progetto, non avete un'anima. Il vostro contratto è un matrimonio di interessi a spese della collettività italiana. Non c'è nulla in questo Documento, come non c'è nulla nei due decreti-legge che da un mese avete approvati, ma che nessuno conosce. Voi stessi avete detto che il decreto sblocca cantieri non sblocca le grandi opere: non sblocca né il TAV, né le 28 grandi opere del Paese e infatti, non produrrà - lo dite voi stessi - alcun beneficio sulla crescita del Paese.

Io lo chiamerei «decreto stagnazione» o «depressione», certificato di un fallimento. Il fallimento lo si vede - lo dico agli amici della Lega - dai dati veri del Paese, Paese, di un Paese che non sogna più perché anche il vostro sogno si è frantumato contro la realtà e l'impotenza di un contratto innaturale, che di fatto ha consegnato il Paese e i Ministeri economici e produttivi a una vecchia sinistra,

che serve chiudere i confini - e siamo d'accordo a chiuderli - se gli italiani fuggono dall'Italia? L'emigrazione è ormai tornata ai livelli degli anni Cinquanta. A che serve fermare gli immigrati - e dobbiamo fermarli - se gli italiani abbandonano il proprio Paese?

*(PD)*. Signor Presidente, autorevoli Ministri, onorevoli senatori, da dove possiamo cominciare? C'è l'imbarazzo della scelta. Seguiamo un criterio cronologico e partiamo dalla serata, dal mio punto di vista infausta, almeno per il Paese, del 27 settembre. quella serata disgraziata, non saprei come altro definirla, il vostro Ministro dello sviluppo economico improvvisò un bel festino, divertendosi alle spalle del nostro Paese e degli italiani, per segnalare due eventi, secondo lui entrambi storici: la fine della povertà nel nostro Paese e una Nota di aggiornamento al DEF, che fissava la crescita all'1,5 per cento.

non si è rivelata una verità e una previsione corretta, ma ciò che riteniamo essere la verità è che lo sapevate perfettamente e stavate dunque mentendo al Parlamento e agli italiani. La povertà, ovviamente, non è stata abolita e anzi, con una certa caparbietà e con determinazione, avete perseguito l'aumento della disoccupazione, che vuol dire povertà povertà economica e morale, perché il nostro Paese ha il diritto di basarsi sul lavoro. La vostra cultura allontana invece il nostro Paese dal lavoro. Oggi, signori Ministri, leggiamo nel DEF che la crescita tendenziale del 2019 sarà dello 0,1 per cento e questo vuol dire una cosa ben precisa: non ci aspetta un cosiddetto anno bellissimo. Non ci aspetta affatto un anno bellissimo, stiamo vivendo un incubo, un periodo di stagnazione, di crescita zero di grandi difficoltà. Il Presidente del Consiglio ebbe però modo di definirlo in questo modo, cercando anche in questo caso, nuovamente, di prendere in giro gli italiani, di raccontare delle fandonie, di far percepire un clima molto lontano dalla realtà. Peggiora il debito, che a dicembre era quantificato in 130,7 miliardi di euro e invece toccherà i 132,6 miliardi Noti bene, si tratta di una vetta storica dal 1924 ad oggi. Che dire, signori Ministri, rappresentanti del Governo? Complimenti al signor Presidente del Consiglio, ai suoi vice: ai suoi vice: ce la state mettendo tutta e ce la state facendo a distruggere il nostro Paese e la nostra economia. PD)*. Torna a salire la disoccupazione. Doveva attestarsi intorno al 10 per cento e toccherà l'11 per cento, nuovamente in crescita dopo anni di riduzione iniziati con il Governo Renzi e rafforzata negli anni dei Governi di centrosinistra. E dire che il suo collega ministro del lavoro Luigi Di Maio aveva la ricetta giusta, la chiamava decreto dignità, la chiave con la quale il Governo gialloverde - il vostro Governo - avrebbe risolto definitivamente non solo la questione già ricordata della povertà, ma anche quella della carenza dei posti di lavoro. Ebbene,

delle imprese, dei risparmiatori, delle famiglie, degli investitori internazionali è crollata grazie alle vostre politiche dissennate. Gli italiani hanno cominciato giustamente - io direi finalmente - a preoccuparsi, hanno rinviato gli acquisti, stanno calando i consumi. Questo è il Paese che voi avete voluto, questa è la condizione generale alla quale voi ci avete portato. Ma come mai sta crollando la fiducia? Tra gli altri motivi, vi voglio ricordare gli argomenti di lite all'interno del Governo, tra i Vice Presidenti del Consiglio, tra i Sottosegretari, tra le maggioranze, viste e riviste nelle interviste televisive, nelle dichiarazioni, nei *tweet* e nei vari modi con i quali voi continuate a parlare al Paese. *(Applausi dal

litigi sulla nostra festa nazionale, quella del 25 aprile, alla quale ci accingiamo ad arrivare con una situazione e con prese di posizione politiche da parte di rappresentanti di questo Governo che sono vergognose. Bisogna andare tutti in piazza a festeggiare la liberazione del nostro Paese. È la nostra festa. Ma non solo, ci sono le direttive del Ministro dell'interno, le ordinanze ai prefetti, e sono rimasto solo agli ultimi momenti di cronaca recente. signor Ministro, cosa succede quando i due principali esponenti di Governo se le danno di santa ragione in ogni occasione utile, e non per grandi motivi ideali,

Signor Ministro, signori Ministri, noi non ci caschiamo. Il Paese l'ha capito, voi fate finta anche su questo, il Governo è uno solo, voi tutti siete responsabili di questo Documento di economia e finanza, voi tutti siete responsabili il Paese è ridotto in queste condizioni. Avete spaventato gli italiani, avete spaventato gli investitori internazionali. Avete fatto crescere lo *spread*. E oggi abbiamo una fotografia impietosa in questo documento. Avete anche rinunciato a dare un messaggio positivo al Paese. Avete rinunciato a dare una ricetta, e indicare una via d'uscita. Non vi vergognate di dire al Paese: qui siamo; qui ci ritroveremo; qui rimarremo; questo è il nostro destino? Questo è quanto avete fatto con questo documento, dove si capisce solo che voi aumenterete le tasse, aumenterete l'IVA e continuerete a impoverire il nostro Paese. E non lo dice il Partito Democratico. Signor Ministro, lo ha detto ieri lei alla Camera. Di fatto, lo dite voi nella vostra risoluzione. Le opposizioni, infatti, possono limitarsi a dire che l'IVA non dovrà aumentare, ma la maggioranza deve dire anche come. Voi avete l'onere del Governo! Avete l'onere delle scelte. Voi avete la responsabilità di aver fatto schizzare il disavanzo del Paese dove è oggi con provvedimenti

Sapete cosa significa aumentare l'IVA? Sapete cosa significa, in termini di consumi? Sapete in che condizioni metterete questo Paese? Ci dovete riflettere. Il Partito Democratico non può accettare questa situazione ma - ahimè il Paese non può accettare questa situazione. Una situazione senza precedenti, con una incapacità di amministrare, di governare, di dialogare, di confrontarsi, di prendere decisioni importanti per il Paese. Io credo che si debba semplicemente dire basta. Il Documento di economia e finanza è la vostra dichiarazione di resa. Vi state arrendendo, ma contro chi? Contro il nemico? No, contro voi stessi, contro la vostra incapacità di governare. Signor Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, dopo un anno (ormai è un anno che state facendo danni), avete messo il Paese in ginocchio. Avete messo in ginocchio l'Italia. Con questo Documento certificate la vostra chiara volontà di dare il colpo di grazia al Paese: bloccate i cantieri, aumentate i disoccupati, create paura e sfiducia negli italiani, aumentate in modo incontrollato il debito pubblico, fate più che raddoppiare lo *spread* a danno del Paese, dei cittadini e delle imprese italiane. Infine riducete a niente la politica estera, non difendete i nostri interessi e, in ultimo, fate anche aumentare l'IVA. Credo sia l'ora di dire basta. Signor Presidente, ringrazio i relatori e tutti i colleghi intervenuti nella discussione per aver reso appassionante, almeno nei toni se non nei contenuti, che qualche volta erano inesistenti o inconferenti, un dibattito che, per un economista, ha pochi motivi di interesse, come mi accingo a spiegare rapidamente ai cittadini che ci ascoltano. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Questo perché il DEF, il Documento di economia e finanza, è solo uno dei tanti atti, il meno significativo, di quella complessa liturgia che va sotto il nome di semestre europeo; liturgia introdotta nel 2010, in piena crisi dei debiti sovrani, con il nobile scopo dichiarato di coordinare le politiche economiche europee ma, in realtà, qualcuno sostiene, per commissariare surrettiziamente i Paesi che erano o che si voleva finissero in crisi. Coordinamento non vi fu e di questo si lamentò il senatore Monti quando, in una nota intervista alla CNN, disse che lui aveva tagliato la domanda interna del Paese, aspettandosi che gli altri facessero crescere la loro. anni dopo stiamo ancora aspettando. Le valutazioni scientifiche su questo strumento di coordinamento sono ancora aperte, ma una cosa è certa: uno degli effetti del semestre europeo è tenerci qui a discutere sul nulla o, peggio ancora, costringere il dibattito sulla politica economica del Paese all'interno di un quadro di riferimento insensato, perché manifestamente fallimentare; quello delle politiche di austerità. Questo quadro di riferimento è fallimentare, come dimostrato dai risultati. Non l'Italia, ma tutta l'Eurozona e tutta l'Unione europea, da quando hanno adottato questo metodo hanno peggiorato la propria *performance* economica in relazione a quella degli altri Paesi dell'economia mondiale. Si tratta di un fenomeno su cui oggi si interroga, senza riuscire a spiegarselo, il Governatore della Banca d'Italia. Eppure, la risposta è sotto i suoi occhi ed è data da politiche di bilancio condannate a essere inadeguate, perché riferite non ai dati economici reali, reali, ma a un concetto evanescente, arbitrario e astratto: il prodotto potenziale, cioè il livello di produzione che un'economia può sostenere senza che l'incremento dell'attività si scarichi in aumento di prezzi. L'insensatezza deriva da qui. Per far contenta l'Unione europea ogni Paese deve assicurare la Commissione di mantenere un tasso di disoccupazione sufficientemente alto, tale da evitare pressioni sui salari. In sostanza, l'Unione europea ci chiede un cospicuo esercito industriale di riserva a garanzia del fatto che i lavoratori - dipendenti, professionisti, commercianti e piccoli imprenditori

tasso di disoccupazione che non accelera l'inflazione. Ma una rosa con un altro nome avrebbe lo stesso profumo e lo stesso vale per un cadavere come questo tipo di coordinamento economico. E allora stiamo parlando del nulla, soprattutto considerando che siamo ben al di sotto di quel tasso di inflazione del 2 per cento che la Banca centrale europea, nel suo insondabile arbitrio, ha indicato come obiettivo di stabilità dei prezzi. Combattere l'inflazione in assenza di inflazione non funziona, ma non ci stupisce da parte di chi combatte il fascismo in assenza di fascismo. PD).* Sono due metodi analoghi per fare la stessa politica di classe a danno degli ultimi, anzi dei penultimi, perché per gli ultimi le risorse si trovano purché non vengano ad abitare ai Parioli. Noi abbiamo voluto invertire la rotta. Ci siamo riusciti? Questa è la domanda. La risposta l'abbiamo avuta dal relatore di minoranza con due parole tombali: fallimento e impotenza; con queste parole ha liquidato la nostra esperienza. l'ultima parte dell'anno precedente è stata caratterizzata da una recessione tecnica, che noi saremmo evidentemente stati impotenti ad affrontare. abbattuto da questa sentenza definitiva, me ne tornavo verso il mio studio, a sorpresa esce un'agenzia della Reuters che certifica che, nel primo trimestre di quest'anno, il Paese ha ricominciato a crescere, come ci ha detto poco fa il ministro Tria. E così abbiamo capito perché il PD parlava di Pillon: per non parlare di PIL, perché se avesse parlato di PIL avrebbe dovuto certificare che quanto stiamo facendo già sta avendo effetti. Allora ragioniamo un attimo sui numeri, anziché su queste previsioni che un quadro di politica particolarmente artefatto ci costringe a produrre. *(Commenti della senatrice Bellanova).* Presidente, desidererei che il mio intervento pacato si svolgesse in un clima

Non è dal DEF (che è non una legge, ma un documento programmatico che risponde a logiche piuttosto particolari) che bisogna valutare l'azione di un Governo, bensì dalla legge di bilancio, che effettivamente dispone i provvedimenti e stanzia le risorse.

sono cambiate. Ci sono i numeri. Tanto per essere chiari, ragioniamo sulla produzione industriale, visto che siamo la seconda potenza manifatturiera europea.

con un incremento che nelle Regioni raggiungeva addirittura l'84,9 per cento. Inoltre, erano anche aumentate le nuove gare, almeno quelle per opere di importo fino a 150.000 euro, dove abbiamo introdotto delle importanti semplificazioni normative: bene, quelle erano aumentate dell'8,6 Questi sono i risultati, e non sono intenzioni ma fatti, e su questi vogliamo essere e saremo giudicati. Un Governo che ha saputo impostare una manovra anticiclica efficace in una fase particolarmente complessa del ciclo economico mondiale

del collega Bagnai non vorrei disturbare i colleghi con il mio intervento. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, nell'aprile del 2018 il Governo Gentiloni Silveri, sconfitto con la sua maggioranza alle elezioni del 4 marzo, presentò un Documento di economia e finanza che si fermava al tendenziale, e lo scrisse in modo esplicito, dicendo: mi fermo al tendenziale, perché giustamente chi ha vinto le elezioni, o comunque il nuovo Governo, dovrà occuparsi delle valutazioni e del programma nazionale di riforma, quindi della parte successiva.

Il DEF è fotografia, è proiezione sul triennio, ma sostanzialmente dovrebbe essere programma nazionale di riforma; dovrebbe essere ciò che sotto il profilo politico il Governo e la maggioranza vogliono fare per il futuro. Nella parte di valutazione fotografica, di valutazione dell'attuale, dopo aver assistito alla Nota di variazioni di ottobre con numeri praticamente da lotto, con una manovra modificata in corso a dicembre, anche con qualche errore rilevante in *Gazzetta Ufficiale*, e costata 100 punti di *spread* che ci stiamo ancora portando dietro oggi

che naturalmente ascriviamo al Ministro dell'economia come merito: una fotografia realistica ancorché amara. Come dichiarato da tutti, abbiamo: un Paese fermo;

discussioni, alimentate nelle nostre Commissioni e in quest'Aula, sui decimali o sullo zero virgola rispetto ai punti di PIL di avanzo Quindi, una manifestazione di disagio economico e sociale, di incertezza e sfiducia. I termini più utilizzati durante le audizioni sono stati quelli di fiducia e sfiducia.

ha parlato di decrescita. Ebbene, ci stiamo avviando alla decrescita felice. La discussione è come coprire il disavanzo, quali tasse aumentare, quali costi tagliare, ognuno con la propria giustificazione; tutto in un quadro legislativo ad oggi invariato, con il risultato automatico (perché è già legge) dell'aumento dell'IVA per 23 miliardi di euro nel 2020 e 29 miliardi nel 2021.

18 miliardi di privatizzazioni, volendo valutare, poi, quali sono e se ci saranno, e, naturalmente, qualche miliardo di debito in più da pagare per i nostri figli.

i giorni di lavoro vengono calcolati dagli statistici in 305: significa 5,8 miliardi al giorno. Basta un giorno di lavoro per fare in modo che lo 0,2 in più diventi 0,1 in meno: un solo giorno lavorativo.

venerdì, a cavallo del sabato, il 28 sabato, il 29 dicembre domenica; l'unico giorno lavorativo, se vogliamo lavorare in pieno, è lunedì 30 dicembre. Pensate quale può essere la conseguenza sulla valutazione della discussione dello 0,2 per cento. Dunque, nel programma nazionale di riforma si doveva dire,

Purtroppo non c'è stata nessuna risposta: totale incertezza. L'IVA è forse sì e forse no, anche nella risposta del Ministro; la *flat tax* è un pezzo sì, ma forse no; i cantieri sì, ma anche no.

il Governo, nel dibattito in Commissione e in Assemblea, ha fatto un lungo elenco di azioni e di provvedimenti, alcuni già attuati, altri messi in cantiere, alcuni approvati oggi dal Consiglio dei ministri:

che le famiglie sono massacrate dalle tasse e dalle tariffe, che le imprese, con il cuneo fiscale attuale, hanno costi sempre più alti mentre, dall'altra parte, i salari sono sempre più bassi. La necessità di una vera riforma fiscale, richiamata anche dal Ministro, significa anche non spezzettare i modelli fiscali, altrimenti si crea davvero confusione. Abbiamo bisogno di riforme che riportino fiducia ed equità sulla società, che è cambiata molto: riforme necessarie, che diano tranquillità, certezze e sicurezza al Paese. questo abbiamo bisogno. Per concludere, onorevole Ministro dell'economia, colleghi, noi tifiamo per l'Italia e appoggeremo qualsiasi misura concreta assunta nell'interesse degli italiani, com'è scritto

Signor Presidente, ci stiamo accingendo a votare il primo DEF del Governo del cambiamento, il Documento di economia e finanza 2019. Abbiamo una situazione internazionale macroeconomica abbastanza complicata: da una parte abbiamo gli Stati Uniti, con i loro dazi; dall'altra, abbiamo la Germania che ha rallentato e abbiamo la Cina, che la fa da padrona e con la quale comunque abbiamo stretto forti rapporti commerciali. quindi una situazione molto complessa, ma in tutto questo iniziamo a registrare dei cambiamenti, dei segnali positivi. Non lo diciamo noi, non lo dice il MoVimento 5 Stelle, lo dice la Banca d'Italia con il bollettino che ha pubblicato oggi. Arrivano segnali positivi su tutto: sulle esportazioni l'andamento è rimasto favorevole; sull'occupazione che è stabile; sulle retribuzioni che sono in crescita. La borsa ha recuperato il 20 per cento dall'inizio dell'anno; anche nel mese di marzo è proseguita la crescita della produzione industriale. Il mercato immobiliare è tornato ai livelli del 2008 per numero di compravendite; gli investitori esteri hanno ripreso ad acquistare titoli di Stato. Un altro segnale di crescita e di cambiamento è arrivato dai cittadini, dai territori, dagli enti locali, grazie alle politiche espansive di questo Governo. *(Applausi dai Gruppi il collega Bagnai e lo ricordo anch'io: nella legge di bilancio sono contenute due misure molto importanti per i Comuni: mi ricollego agli avanzi di gestione, che sono stati sbloccati, e mi ricollego ai famosi 400 milioni che i Comuni hanno iniziato a spendere. Grazie anche a queste misure

hanno tolto risorse, ma hanno lasciato numerosi compiti da svolgere alle Province: noi stiamo "mettendo le pezze", piano piano, perché non abbiamo la bacchetta magica e su questo riusciamo ad ottenere segnali positivi dalle persone, dai cittadini e dagli stessi enti locali che hanno oggi più fiducia nell'amministrazione centrale dopo anni

ci saranno 100.000 famiglie nelle quali almeno una persona tirerà un sospiro di sollievo: una persona che ha lavorato almeno trentotto anni, pagando i contributi previdenziali all'INPS, ed è arrivata all'età di sessantadue anni. Ebbene, queste famiglie potranno avere una persona che potrà dedicarsi agli affetti, alla famiglia, ai nipoti, agli *hobby*, e farà una cosa indispensabile per il nostro Paese, ovvero lasciare un posto libero che verrà sicuramente occupato da qualcuno più giovane. Presidente, sono segnali importanti. Sappiamo benissimo che, secondo i nostri detrattori, le statistiche dicono cose diverse, perché queste misure hanno un impatto diretto sull'occupazione e sulla disoccupazione, ma sappiamo anche che si tratta di statistiche che non tengono conto del fatto che i dati cambieranno da qui a breve.

Mi spiace ammetterlo, ma queste famiglie adesso potranno consumare con più facilità e porteranno anche un incremento alla nostra economia, che, purtroppo, per troppi anni è stata dimenticata. Presidente, andiamo avanti perché segnali di ottimismo arriveranno anche dopo Pasqua con l'approvazione del decreto crescita e del decreto sblocca cantieri, che daranno una mano al settore delle costruzioni, un settore fondamentale, trainante per la nostra economia. Anche da lì avremo risultati concreti,

noi, Presidente, siamo più "schisci", stiamo più con i piedi per terra. Presidente, sull'avanzo primario, chi ci ha preceduto nel 2013 stimava a un anno e a tre anni un avanzo del 2,4 e del 4,7; che cosa si è realizzato? Un 1,9 e un 1,4. Era il Governo Letta. Poi è arrivato il Governo Renzi: nel 2015 ha previsto 1,7 e 4,3; che cosa si è realizzato? Un 1,5 e un 1,6. Presidente, è ora di dire basta a queste fantomatiche stime che non stanno in piedi. Presidente, noi prevediamo un umile 1,2 per quest'anno e un altrettanto umile 2,0 per l'anno prossimo, che sicuramente riusciremo a realizzare.

che sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Patuanelli e Romeo, accettata dal Governo, sono stati presentati 15 emendamenti, i cui testi sono in distribuzione.

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione della situazione in Libia». Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte. Gentile Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, accolgo con piacere la richiesta di illustrare anche a questa Aula lo stato della situazione libica, sulla quale ho già riferito alla Camera dei deputati la scorsa settimana. Gli ultimi sviluppi in Libia, in particolare l'*escalation* militare, continuano ad essere motivo di forte preoccupazione per l'Italia, per l'Europa e per la comunità internazionale intera. La cornice di sicurezza del Paese rimane estremamente fragile e fluida, a seguito dell'avvio, lo scorso 3 aprile, dell'offensiva militare dell'LNA verso Tripoli, sulla scia della conquista, a inizio dicembre, di importanti aree del Sud del Paese, con l'obiettivo dichiarato di combattere il terrorismo e stabilizzare la regione. Il 6 aprile il presidente del governo di accordo nazionale al-Sarraj ha inviato un messaggio televisivo alla nazione, nel quale ha espresso sorpresa per l'aggressione posta in essere nel corso delle trattative in vista della Conferenza nazionale e ha assicurato una ferma risposta a quello che ha definito un tentato colpo di Stato. Con il passare dei giorni, gli scontri sono proseguiti con alterne vicende, in un quadro di sostanziale equilibrio tra le forze in campo. I principali quadranti di scontro si collocano al momento a Sud della capitale, dove si concentra la resistenza delle forze facenti capo al Governo di accordo nazionale contro l'avanzata dell'LNA, e ad al-Jufrah, dove sono attive le forze di Misurata, con l'obiettivo di compromettere la lunga catena logistica e di rifornimento dello stesso autoproclamatosi esercito nazionale libico. Ad esacerbare ulteriormente il livello dello scontro, in particolare nelle giornate del 16 e del 17 aprile scorso, si è verificato un prolungato lancio di razzi Grad da parte di unità dell'LNA verso diverse zone della città di Tripoli, che ha provocato anche alcune vittime tra la popolazione civile. Si registra un aumento delle tensioni anche nell'area di Sirte, stati preposizionamenti delle forze misuratine e la dichiarazione, da parte dell'LNA, dell'avvio di un'operazione nell'area. Lo stallo sul terreno, in ragione dell'apparente parità delle forze in campo, ha dunque inevitabilmente determinato un'evidente *escalation* militare, con un crescente uso di armamenti più potenti e di artiglieria pesante e un ricorso sempre più frequente all'aviazione da parte di entrambe le parti. Ad oggi gli scontri hanno spinto circa 18.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni e gli sfollati interni sembrerebbero ancora in aumento. La stima esatta delle vittime e dei feriti, al momento alcune centinaia, non è certa, stante la difficoltà di conciliare le informazioni ufficiali con quelle ricevute dal terreno. Anche la missione dell'ONU condivide comunque la percezione di un probabile aggravarsi della crisi. In questa prospettiva e in questa situazione il rischio di una crisi umanitaria è concreto. La situazione di caos e violenza accresce fortemente anche il rischio di una recrudescenza del fenomeno terroristico, del resto ancora ben presente in Libia, come confermato dall'attentato compiuto il 9 aprile da Daesh a Fuqaha (al-Jufrah) e come dimostrato dalle infiltrazioni di elementi jihadisti tra le fila di milizie e gruppi combattenti. Il contrasto al terrorismo e al flusso di *foreign fighter*, anche in ragione dell'evoluzione del quadrante di Siraq, rimane dunque una delle principali sfide con cui il Paese e l'intera comunità internazionale devono responsabilmente confrontarsi. Per quanto riguarda le possibili conseguenze sui flussi migratori verso l'Italia o altro territorio sempre dell'Unione europea, al momento, al di là delle cifre circolate nei giorni scorsi (anche a fini propagandistici), dalle informazioni in nostro possesso non emerge un quadro di imminente pericolo. Su tutto questo complesso quadro di sicurezza manteniamo naturalmente molto molto alta la nostra attenzione anche attraverso la nostra sede diplomatica e i servizi di *intelligence*. È, però, evidente che in una situazione di tale fragilità non ci sia tempo da perdere. Il protrarsi del conflitto, che potrebbe degenerare in una vera e propria guerra civile, va scongiurato rapidamente e con tutto l'impegno politico necessario. Sul piano politico gli sviluppi sul terreno, per molti versi inattesi soprattutto nella loro rapidità, hanno inevitabilmente determinato l'insuccesso della missione del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres il rinvio della Conferenza nazionale che - vi ricordo - era programmata per il 14 e 16 aprile a Gadames. È palese, del resto, che alla base di questa nuova crisi vi sia anche la perdita di coesione della comunità internazionale, che non è riuscita a offrire evidentemente indicazioni univoche nell'assicurare soprattutto con piena compattezza il proprio sostegno all'azione delle Nazioni Unite, come invece era riuscita a fare anche in occasione della Conferenza di Palermo. È sul ritorno a questa questione che stiamo, dunque, profondendo le nostre energie e spendendo il nostro peso politico. Come ricordato dallo stesso Guterres nel suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 aprile, l'involuzione in atto non ci deve infatti far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica, che è l'unica davvero sostenibile. Certamente l'obiettivo principale e immediato in questa fase continua a essere la cessazione delle ostilità e l'instaurazione di una tregua che permetta innanzitutto di proteggere la popolazione, gestire gli aiuti e favorire la ricostruzione di un clima di fiducia necessario per sedersi nuovamente al tavolo dei negoziati. Sono stati effettuati dei tentativi di mediazione da parte del rappresentante speciale dell'ONU Ghassan Salamé finalizzati al raggiungimento di un accordo tra le parti per il cessate il fuoco e la possibile ripresa del confronto negoziale. La maggiore difficoltà su questo versante viene dalle condizioni che le parti intendono imporre per un ritorno al tavolo della diplomazia. Sin dall'inizio della crisi, l'Italia ha condotto un'intensa attività diplomatica a più livelli e a tutto campo. Un'attività che si è rivolta alle parti libiche, ai principali attori regionali e internazionali, ha coinvolto le Nazioni Unite e l'Unione europea, al fine di scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione sul terreno, che potrebbe avere gravi conseguenze per la popolazione libica e la stabilità dell'intera regione euro mediterranea. Su impulso italiano il 5 aprile scorso i Ministri degli esteri dei Paesi del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Libia che ben fotografa la nostra posizione. I Ministri hanno, in particolare, riaffermato che non esiste una soluzione militare al conflitto libico; hanno reiterato il pieno sostegno al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e al suo rappresentante speciale Salamé per trovare una soluzione allo stallo politico in vista di elezioni credibili e pacifiche, in linea con quanto convenuto a Palermo. Hanno fatto appello a tutti i libici affinché sostengano costruttivamente il processo onusiano e hanno invitato la comunità internazionale a mostrare piena coesione in vista del comune obiettivo della stabilizzazione della Libia. Abbiamo giocato, inoltre, un ruolo chiave nell'elaborazione della dichiarazione dello scorso 11 aprile dell'alto rappresentante Mogherini per conto dell'Unione europea sulla situazione in Libia, anch'essa pienamente in linea con la posizione italiana. Come ho avuto modo anche di ricordare la scorsa settimana dinanzi alla Camera dei deputati, in questi mesi, ma anche in questi giorni e in queste ore sono stato in contatto diretto con i due principali attori libici,

Frequenti sono anche i contatti degli altri Ministri del Governo, a partire naturalmente dal ministro Moavero Milanesi, in un quadro di coordinamento, assicurato dalla cabina di regia, che all'indomani dello scoppio della crisi ho costituito a Palazzo Chigi. A tutti i nostri interlocutori abbiamo manifestato la nostra forte preoccupazione per l'*escalation* militare e per i rischi di una crisi umanitaria, nonché l'urgenza di lavorare in direzione di un cessate il fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare, preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio. Si tratta, come detto, di una strada obbligata per ridare spazio al dialogo politico e ricostruire un minimo di fiducia tra le parti, ai fini di un processo credibile e sostenibile. È evidente che favorire il cessate il fuoco e la ripresa del dialogo politico non può prescindere dalla disponibilità delle parti ed è per questa ragione che crediamo in un approccio inclusivo che, nel rispetto del diritto internazionale, attraverso un'azione di equilibrata mediazione, possa mantenere aperto il canale di dialogo tra le parti e dare ascolto alle legittime aspettative del popolo libico, estenuato da otto anni di instabilità e di insicurezza. Il nostro sostegno al Governo di accordo nazionale, infatti, è andato in questi mesi di pari passo con una forte azione di *moral suasion*, volta ad identificare ogni possibile spazio di intesa politica con gli altri attori, a partire naturalmente dal riconoscimento del ruolo del generale Haftar, non solo in Cirenaica, ma anche sul piano nazionale. A questo mi sono dedicato in particolare nel mio incontro con al-Sarraj, a margine del vertice tra Unione europea e Lega araba, che si è tenuto a Sharm el-Sheikh a fine febbraio, proprio alla vigilia dei colloqui di Abu Dhabi, che pure avevano acceso la fiamma della speranza, perché si erano svolti al fine di ragionare su un possibile specifico accordo tra le parti. A questo continuo a dedicarmi, nella consapevolezza che gli spazi di manovra attuali sono certo esigui, ma anche con la certezza che non vi sono alternative credibili e sostenibili. Come osservavo in precedenza, questa crisi è frutto certamente di debolezze che definirei strutturali del contesto locale, ma anche di influenze esterne, che non sempre sono andate nella direzione della stabilizzazione. L'instabilità protrattasi per otto anni in Libia va del resto inserita in un contesto regionale, che appare non meno critico e che dobbiamo assolutamente preservare. Si pensi ad esempio ai più recenti sviluppi in Algeria, ai rischi di ripercussioni sulla Tunisia e agli sviluppi sul quadrante mediorientale. L'obiettivo di favorire il recupero di una più ampia coesione internazionale sul *dossier* libico è dunque oggi più indispensabile che mai e mi spinge ad un intenso impegno sul piano diplomatico, anche attraverso le mie numerose missioni all'estero. Con tutti i Ministeri interessati, col mio *staff* diplomatico e i competenti organismi stiamo ulteriormente rafforzando il filo diretto con i principali *stakeholder* internazionali, a partire dagli Stati Uniti, dai *partner* europei e dagli attori regionali più influenti in Libia. Particolarmente intensa è l'interlocuzione con Washington. Come è noto è stato anche diffuso a mezzo stampa - ho avuto ieri un colloquio telefonico con il presidente Trump, con cui abbiamo condiviso la preoccupazione per l'*escalation* militare e per i rischi di una crisi umanitaria. il presidente Trump abbiamo concordato di restare in stretto e diretto contatto sin dai prossimi giorni, dalla prossima settimana, per individuare una soluzione sostenibile alla crisi libica e quindi perseguire una soluzione politica. Nei giorni scorsi ho avuto uno scambio di valutazioni con la cancelliera Merkel, che come me e con me ritiene imprescindibile e urgente la cessazione delle ostilità e il riavvio del dialogo ai fini di una soluzione politica. In più occasioni ho discusso anche il *dossier* libico con il presidente Macron, da ultimo a Bruxelles. Rimaniamo in stretto contatto anche a livello di *staff*, con l'obiettivo comune di perseguire la stabilità e lo sviluppo della Libia. Una Libia instabile, del resto, non può soddisfare alcun interesse nazionale di nessun Paese. Divergenze sul tema non solo appaiono illogiche, ma soprattutto appaiono inammissibili. Stretto il raccordo anche con i *partner* della regione per ottenerne un coinvolgimento il più possibile lineare rispetto al processo politico che prefiguriamo e che stiamo perseguendo. Dal Qatar all'Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti alla Turchia, passando per Tunisia e Algeria, il confronto è aperto e costante con tutti. Oltre a questa intensa attività politico-diplomatica e nonostante la gravità degli scontri in corso, l'Italia continua ad essere presente sul terreno. La nostra ambasciata a Tripoli ad oggi è pienamente operativa, il personale militare italiano presente in Libia - prevalentemente concentrato a sostegno dell'attività dell'ospedale di Misurata e della Guardia costiera libica - non è stato evacuato. A tutti loro vanno il nostro plauso e la nostra ammirazione per l'impegno e la dedizione con cui assolvono il proprio compito anche in condizioni di oggettiva criticità. Monitoriamo costantemente le condizioni di sicurezza, ma finché queste ultime lo consentiranno, siamo intenzionati a rimanere a fianco del popolo libico e siamo intenzionati a continuare a lavorare in prima linea per assicurare una transizione sostenibile, forti del nostro approccio improntato al massimo rispetto per la popolazione libica e forti di un senso di responsabilità che, se mi consentite, si acuisce di ora in ora, perché ci deriva dal fatto - direi oggettivo - che siamo tra i pochi Paesi stranieri che hanno una credibilità che ci pone in condizione di interloquire con tutti gli attori libici. L'Italia recentemente ha aderito alla richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità per la fornitura a scopi umanitari di *kit* sanitari in Libia. La fornitura consentirà all'Organizzazione mondiale della sanità di proseguire il programma di distribuzione dei medicinali e di poter disporre di attrezzature medico-sanitarie per le prestazioni mediche *in loco*. La fornitura sarà disposta dal deposito umanitario di Brindisi e consegnata, tramite l'ambasciata a Tripoli, al Ministero della salute libico. Abbiamo inoltre già dato la nostra disponibilità ad entrambe le parti per assicurare l'assistenza sanitaria italiana per la cura dei feriti provenienti da entrambi gli schieramenti a causa degli scontri delle ultime settimane stiamo valutando - ma si tratta veramente delle ultimissime ore - anche la possibilità di rinforzare il nostro presidio medico dell'ospedale di Misurata. Sui corridoi umanitari nella regione, il nostro Paese, dai tempi della primavera araba ad oggi, ha mostrato - mi sia consentita questa espressione - il miglior volto dell'Europa.

e c'è stata anche qualche nota critica sulla presunta scarsa incisività dell'azione italiana. In realtà - e lo osservavo anche alla Camera - la tempistica degli scontri ci induce a pensare che stessimo procedendo nella giusta direzione e che si è quindi voluto deliberatamente far deragliare un processo politico concreto e ben avviato. Dobbiamo quindi profondere ogni energia nel tentativo di recuperarlo, evitando che ancora una volta possano prevalere in Libia le forze dell'instabilità permanente, della violenza, della conservazione di uno *status quo* di cui il popolo libico è il primo a pagare le spese. Ancora, ho più volte parlato di ricostruzione della fiducia tra le parti e di riavvio del percorso negoziale per individuare una soluzione sostenibile e ho richiamato il principio che ha sempre ispirato la nostra azione di Governo: quello di inclusività. Sin dalla conferenza di Palermo, abbiamo basato la nostra azione sulla necessità di coltivare e alimentare un dialogo tra tutte le diverse anime politiche libiche, nella consapevolezza della complessità di quella realtà. Ancora, «inclusività» non significa - tengo a sottolinearlo - ambiguità o indecisione, bensì coerenza con un approccio che parte proprio dalla considerazione dei nostri interessi strategici e, quindi, dall'esigenza di garantire la stabilità della Libia. Significa anche equilibrio, visione e mantenimento di una capacità di mediazione che è essenziale poter esercitare per far tacere le armi e far parlare la politica. È illusorio e pericoloso perseguire una soluzione che punti a imporre con la forza le ragioni di alcune fazioni e di alcuni Paesi nei confronti degli altri. osservato, infine, alla Camera e tengo a ribadirlo qui, che non ci sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare scorciatoie militari e, in ultima analisi, il rischio di una guerra civile in Libia. Come purtroppo i fatti stanno dimostrando, la violenza genera violenza e non serve né gli interessi della popolazione, che già risulta, allo stato, colpita o addirittura sfollata né quelli della comunità internazionale né, certamente, quelli dell'Italia. *(Applausi dai

come succede molto raramente, non sarà in diretta su Radio Radicale. E non lo sarà perché, per un giorno, forse due, Radio Radicale ha deciso di dedicare tutto lo spazio programmato all'approfondimento e al ricordo di Massimo Bordin. Però, signor Presidente, essa è dovutamente registrata, sarà dovutamente archiviata in quel gioiello che è l'archivio di Radio Radicale e potrà essere ascoltata nei prossimi giorni o nei prossimi anni.

Fate una gara: non c'è problema. Anzi, l'abbiamo chiesta ogni anno. Vede, privatizzare l'archivio di Radio Radicale non è proprio possibile. Lei lo sa meglio di me. Non mi dilungo,

a volte, sia segno di forza e non di debolezza. Diceva Sciascia: «contraddissi e mi contraddico» e ne vado orgoglioso. Detto questo, vengo brevemente alla Libia. alla Libia. Signor Presidente del Consiglio, io immagino che tutte le cancellerie siano all'opera, soprattutto, intanto, per evitare l'esplosione di una guerra civile e una crisi umanitaria, evidentemente. Direi, però, che questo è un po' un modo di dire. Non mi pare, infatti, che tutte le cancellerie dialoghino nella stessa direzione. Per non aggravare l'imbarazzo non farò nomi, ma non so se sia giusta la voce, che mi è appena arrivata, della rottura delle relazioni diplomatiche tra al-Sarraj e la Francia.

appunto, questi tre conflitti, uno intralibico, uno intramusulmano (con il Qatar e la Turchia, da una parte, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi uniti dall'altra parte) e uno internazionale

E se c'è un'altra ragione per cui abbiamo bisogno di più Europa e di superare il blocco dell'unanimità del Consiglio e dei vertici di Capi di Stato, non dobbiamo guardare molto lontano. Guardiamo alla Libia, con i rischi che lei giustamente sottolineava, di contagio con la Tunisia, con una situazione men che stabile in Algeria e un'altra situazione più esplosiva (basta guardare una mappa) nel Sudan.

perché, se ho capito bene, non ci sono più navi, ma solo gli aerei, per fare cosa non si è capito. E non è ovviamente impensabile che la gente scappi dalla guerra, in particolare da quella civile.

Quindi, lo sforzo diplomatico è l'unico che abbiamo davanti. Poi avremo tempo di guardare indietro, vedere cosa è successo, chi ha sbagliato, eccetera. Ma Ma oggi abbiamo questa responsabilità, per la parte che ci riguarda, rispetto soprattutto alla popolazione libica. Aspettando

Non c'è altra scelta. Quanto al Sudan, al-Bashir deve andare alla Corte penale internazionale. Questa è l'unica via possibile per evitare ulteriore spargimento di sangue. la prego di seguire con grande attenzione questa iniziativa e possibilità.

sulla situazione che si sta verificando alle porte di casa nostra, al confine meridionale dell'Italia, nel Paese in cui vi è il nostro prioritario interesse strategico: la Libia. Il Primo Ministro ha parlato di una crisi umanitaria che rischia di destabilizzare l'intero Mediterraneo. La Libia rischia di diventare la nuova Siria, in una guerra civile, per procura, tra potenze sunnite, in cui l'Europa - non solo l'Italia - non avrà più voce. Ci chiediamo anzitutto come mai questo sia accaduto così velocemente negli ultimi mesi rispetto al clima e all'immagine che lei, presidente Conte, aveva dato a Palermo il 13 e 14 novembre scorso. Come mai la situazione è degenerata e se si poteva evitare che degenerasse. Tutti sapevamo che il comandante Haftar si era mosso dalla Cirenaica aiutato da due potenze imperiali europee e da potenze sunnite nel Sud del Paese, conquistando anche i pozzi petroliferi dell'ENI.

e ha diviso le sue alleanze internazionali. In questo contesto, il nostro Governo, consapevole di quello che stava accadendo nel principale Paese di interesse strategico dell'Italia,

rendendo afono il Ministro degli affari esteri, che non è nemmeno presente in quest'Aula accanto a lei. Ciò al punto che lei è stato costretto ad accentrare tutti i poteri e tutta la rappresentanza a Palazzo Chigi ed ha fatto bene. Il Governo si è anche diviso dai suoi alleati internazionali. Aveva ottenuto da Trump nel primo colloquio a Washington una sorta di protezione sui nostri interessi in Libia. Nel frattempo, ci siamo divisi dagli Stati Uniti su Venezuela, ci siamo divisi dagli Stati Uniti sulla Cina e in maniera avventata abbiamo annunciato il ritiro dall'Afghanistan. Nel contempo ci siamo isolati in Europa; nel contempo siamo apparsi strani alla Russia, a cui avevamo promesso addirittura che ritirassimo le sanzioni; nel contempo abbiamo messo un dito nell'occhio ad al-Sisi; nel contempo abbiamo attaccato la Turchia di Erdogan. Non so se sia stata una politica saggia quella di dividersi e dividerci rispetto al nostro contesto internazionale, mentre era in palio proprio la Libia, Paese per noi prioritario. presidente Conte, noi parliamo a tutti, certo: l'Italia è l'Italia, soprattutto in Libia e nel Mediterraneo; ma temo che non ci ascolti più nessuno. Libia e nel Mediterraneo; ma temo che non ci ascolti più nessuno. E anche le indiscrezioni che sono uscite ieri dal colloquio che lei ha finalmente avuto col presidente Trump sono inquietanti, perché mettere sullo stesso podio, nello stesso colloquio telefonico, il Venezuela e la Libia ci fa capire qualcosa, chi conosce questo Paese e la sua politica estera. Cosa dobbiamo fare? Esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto in questi mesi. Innanzitutto, ci vuole l'unità del Governo. Non è ammissibile che vi siano dichiarazioni difformi da campagna elettorale in un Governo che è alla guida di un Paese, l'Italia, che rischia di subire la più grave sconfitta della sua storia repubblicana, pregiudicando i propri interessi al punto da rischiare una crisi umanitaria, politica, economica, emergenziale alle sue porte, in Libia. Non sono ammissibili divisioni nel Governo. Dico di più. Lei dovrebbe fare appello all'unità del Paese, perché quello che noi rischiamo è davvero troppo rispetto a quello che il Governo ha messo in campo. In questi momenti è assolutamente necessario esprimere la massima unità nazionale. Poi giudicheremo l'operato del Governo, ma oggi occorre agire in fretta per recuperare quello che non si è fatto in questi mesi, in cui si è passati dalla foto idilliaca di Palermo, in cui l'Italia era tornata in campo, al punto in cui in Libia non c'è più l'Italia, non ci sarà più l'Europa, ma ci sarà una guerra civile tra potenze sunnite fondamentaliste che alimentano il terrorismo islamico.

La Libia è di fronte all'Italia; è interesse nazionale, non solo per l'Italia, come ha ricordato lei, ma soprattutto per l'Italia; che la Libia sia stabile è fondamentale per noi non solo per gli approvvigionamenti energetici: pensiamo a cosa potrebbe voler dire per l'Italia il rischio di una catastrofe umanitaria. Tripoli è una città di due milioni di abitanti, un terzo degli abitanti della Libia; che cosa potrebbe succedere, se scoppiasse davvero una guerra civile? Relativamente a questo, come conseguenza, vi è il rischio di un riacutizzarsi delle crisi migratorie.

ma, dopo due o tre anni di fragile equilibrio, la situazione si sta sgretolando. Non riteniamo certo il Governo responsabile della crisi - ci mancherebbe altro - però mi permetto di muoverle qualche appunto. Un'eccessiva enfasi sui risultati della Conferenza di Palermo: si è parlato di un protagonismo risolutivo dell'Italia, ma purtroppo non è stato così. Anche rispetto ad Haftar, forse sono stati un po' troppi i tappeti rossi lanciati davanti a lui; era giusto invitarlo, ma Nel frattempo, però, il *dossier* non veniva maneggiato con la cura e la continuità necessarie. necessarie. Non si è più investito nella lotta ai trafficanti, come ricordava la senatrice Bonino: la missione Sophia, che era così importante, è una missione marittima che adesso non ha più navi in mare e l'Italia non l'ha sostenuta. Ma anche sui corridoi umanitari si poteva lavorare per una migrazione regolare; anche su quello non si sono fatti molti passi avanti. poi, è risultata essere sempre più isolata. Punti di vista e opzioni diverse rispetto alla Francia li conosciamo, ma proprio per questo si richiedeva un lavoro più forte con l'Unione europea. Lei oggi ha detto che con la Germania abbiamo gli stessi punti di vista, ma in questi mesi avremmo dovuto lavorarci di più

Anche per rinsaldare il dialogo europeo, forse le parole così ruvide che spesso il ministro Salvini ha usato nei confronti di Juncker o la foto *opportunity* con i *gilet* gialli che ha fatto il vice *premier* Di Maio non sono stati proprio un viatico per migliorare i nostri rapporti. Lei ha parlato della cabina di regia. Giusto che sia a Palazzo Chigi e giusto che lei ci lavori direttamente; ma per farla funzionare penso le servirebbe anche un semaforo per dirigere il traffico fra le dichiarazioni contraddittorie e qualche segnale di *stop* ai suoi Ministri. Assistiamo, infatti, con preoccupazione a una rissa continua fra i Ministri e fra gli azionisti di maggioranza della sua coalizione:

la manda anche alla Marina, tanto la ritiene fondamentale, anche se la Marina dipende dal Ministero della difesa; ma Di Maio dice che non è con una direttiva che si fermano tutti i migranti che potrebbero arrivare. L'interesse nazionale dovrebbe spingere tutto il Governo a lavorare accanto ai diplomatici, ai militari, all'*intelligence* (lei ha ricordato che sono sul campo, a Tripoli, a Bengasi, a Misurata), non a usare strumentalmente corpi dello Stato per scontri da campagna elettorale. Ministri che non si parlano, che si attaccano sui giornali; stati maggiori che sono costretti a ribadire che non possono essere tirati per la giacchetta da nessuna parte

allora, e la prego di lavorare in questo senso: riporti dritta la barra del Governo; quella libica è una questione troppo importante. Lei lo ha detto: non va avallata l'offensiva di Haftar; va scongiurato che il conflitto diventi una guerra civile, e su questo le diamo piena ragione e appoggio. Bisogna provare a far ripartire il lavoro che era stato fatto dall'ONU per preparare la Conferenza nazionale sulla Libia. Bisogna coinvolgere di più l'Unione europea e gli Stati Uniti, - la prego - tenendo lontano questo *dossier* dalla campagna elettorale. Su questo fronte lei avrà il nostro sostegno perché l'Italia sulla questione libica deve essere unita. Signor Presidente, innanzi tutto voglio ringraziare il nostro Presidente del Consiglio per la disamina odierna e per l'azione di questo Governo nel contesto della crisi libica. Vorrei ricordare che la crisi in Libia non è cominciata questo mese né è iniziata nel 2018, ma nel 2011, per le colpevoli - a mio avviso iniziative militari di una potenza europea, seguita, purtroppo, dalle altre. Questo Governo ha il merito di aver tracciato una linea, che è quella di realismo, dicendo che l'anticamera a Sud del nostro Paese non può essere lasciata passivamente alle azioni di altri. Con equilibrio, perseveranza e pazienza il nostro Governo è riuscito a intavolare un'azione diplomatica che ha portato alla Conferenza di Palermo alla fine dello scorso anno. Il tentativo di *Blitzkrieg* da parte di Haftar nella parte occidentale della città di Tripoli non è andato come lo stesso sperava, avendo cercato di alterare *manu militari* - stile vecchia politica di potenza - il quadro di prospettiva di una soluzione diplomatica (la conferenza dell'ONU per portare a nuove elezioni il Paese era programmata per la settimana successiva a quella dell'attacco). il Governo ha avuto il merito di riportare all'attenzione dello scenario internazionale l'Italia come protagonista della politica del Mediterraneo meridionale. Non abbiamo più accettato passivamente i flussi di immigrati che venivano riversati dalle mafie internazionali sulle nostre coste; non abbiamo più accettato passivamente l'intervento di potenze che si qualificano, nei fatti, come *competitor* o addirittura avversari del nostro Paese,

*in primis*, la protezione delle infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas destinati al nostro Paese; *in secundis* - e solo in ordine di esposizione - il pericolo di una crisi umanitaria incontrollata infiltrata da elementi terroristi jihadisti. Infatti, se nel Nord della Libia si combatte, nella Regione sahariana del Fezzan, Isis, Daesh e Al Qaeda sono ritornati operativi tentando di consolidarsi a livello territoriale occupando piccoli paesi e villaggi, ma che in una zona con scarse comunicazioni sono fondamentali. Al pericolo dei terroristi infiltrati che arrivano in Europa si può aggiungere il pericolo di destabilizzazione con un rinnovato Stato islamico, questa volta in Libia, o una rinnovata Al Qaeda non nelle grotte dell'Afghanistan ma in un qualche oasi remota del deserto. Ringrazio il nostro Presidente del Consiglio per l'azione. Potrei chiedere di appellarsi all'Unione europea, ma la cosa mi fa un po' preoccupare visto che, una volta di più sulla crisi libica,

e di conseguenza non è lì che potremmo trovare appoggio per una soluzione diplomatica e di civiltà per il popolo libico e per la stabilità dell'Italia e dell'Europa. Rimangono le Nazioni Unite: Rimangono le Nazioni Unite: mi aspetto una voce forte dell'Italia in seno a tutti gli organi dell'ONU, perché è l'unica strada per arrivare a una soluzione diplomatica; diversamente, non avremo la possibilità

la stabilizzazione è necessaria perché lì avvenga il controllo di queste masse, tra le quali non si nascondono rifugiati, ma migranti economici e soprattutto, a volte, non migranti semplici delinquenti. Preservare gli interessi nazionali, a volte, vuol dire andare oltre i confini nazionali. Su questo punto concludo ringraziandola, signor Presidente del Consiglio, perché ha il nostro supporto e la nostra fiducia per quello che ha fatto e per quello che farà.

Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il quadro libico ci restituisce ora dopo ora uno scenario sempre più inquietante. Ai nostri confini si consuma una guerra civile che assume su di sé conflitti e contraddizioni internazionali, regionali e financo religiosi, con una partita tutta interna al mondo sunnita. Il rischio che la Libia diventi una nuova Siria o un nuovo Yemen, se non anche peggio, è più che una mera ipotesi. A questo, come sappiamo, contribuisce l'irresponsabilità di molti attori interni ed esterni al Paese. Del resto, la dicono lunga le divisioni che albergano all'interno di tutti gli organismi internazionali, dal Consiglio di sicurezza, alla Lega Araba, passando per l'Unione europea. Dobbiamo sapere però che, se non ci sarà accordo tra le potenze in campo, non ci sarà soluzione possibile. Proprio il campo europeo è quello che più ci interessa da vicino, ma non nascondiamoci dietro dichiarazioni di facciata, ipocrite e inutili: c'è un conflitto tra noi e la Francia di ordine politico, economico e direi anche di visione geopolitica del Mediterraneo. Non è una novità, certo, ma dobbiamo dirci la verità: se non lo facciamo e usiamo toni trionfalistici come a Palermo lo scorso novembre, dove già si vedeva arrivare la crisi libica di questi giorni, visto che erano già in corso le operazioni politiche militari di Haftar nel Sud del Paese, difficilmente avremo una posizione nazionale forte, chiara e sostenibile, non soggetta agli umori della maggioranza e dei conflitti politici, che non dovrebbero mai e poi mai interessare la politica estera di un Paese serio. Qualcuno chiama questa responsabilità; mio padre la chiamava interesse nazionale; io, più prosaicamente, la chiamo serietà. Detto ciò, ci spiace ravvisare che lo sviluppo di una posizione italiana sulla Libia non sfugga, non allo scontro prevedibile tra maggioranza e minoranza parlamentare, ma addirittura a quello interno alla maggioranza e al Governo. In questi giorni e in queste ore parlate con più e troppe voci: non si capisce in capo a chi stia la conduzione della politica estera e quale linea o strategia si intenda seguire. Credetemi, non è certo il miglior modo per vincere sui francesi - ammesso che, come qualcuno di voi pensa, si tratti di un *derby* con i cugini d'oltralpe - né per trovare una soluzione. Il conflitto è più serio e largo: più serio, perché in ballo c'è la nostra funzione nel Mediterraneo, l'unico spazio per avere una proiezione geopolitica e geoeconomica internazionale; più largo, poiché si stanno disegnando sulla partita libica nuove alleanze. E noi con chi stiamo? Allo stato, appaiamo isolati: nessuna Nazione europea ci segue; invochiamo l'aiuto degli Stati Uniti, ma poi firmiamo i *memorandum* con i cinesi e pasticciamo sul Venezuela. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. È vero che qualcuno in Libia gioca sottobanco alla guerra, mentre recita pubblicamente il il copione del buon pacifista, ma attenzione a non far interpretare all'Italia la parte dell'apprendista stregone. Non ho capito, signor presidente Conte, che ruolo immaginate per l'Italia nel conflitto libico (e lo dico con preoccupazione, senza polemica). Siamo forza di dialogo tra le parti, come credo dovremmo essere, o partigiani degli uni che non vogliono scontentare gli altri, ottenendo il risultato di scontentare gli uni e gli altri? Ci facciamo tirare la giacca da Maitig, facendoci dire dalle colonne dei quotidiani cosa dobbiamo fare; lo stesso che nei mesi scorsi ha lavorato per indebolire il già precario al-Sarraj. Ci facciamo dettare la linea dai quatarini, diventando una sorta di alleati dei Fratelli musulmani, oppure proviamo a stilare e a suggerire noi un'agenda per la tregua? Vogliamo fermare i rifornimenti di armi ad Haftar o pensiamo di armare sottobanco Tripoli, come qualcuno va vociferando? Fate un gran parlare di strategie, ma di strategico vedo solo il gran parlare che se ne fa. Se qualcuno pensa che il nostro interesse è fare qualche accordo con qualche milizia libica che gira in Italia a buon mercato, ecco, io penso che commetteremmo nuovamente gli stessi errori del recente passato. Attenzione quindi a giocare con il fuoco. Se, passata questa offensiva di Haftar, la vostra idea è quella di sostituire il debole al-Sarraj con qualche altro esponente a noi caro commetteremmo un grande errore. Infine - e concludo - attenzione alla minaccia terroristica. Entrambi le parti libiche si accusano l'un l'altra di favorire il ritorno di un'offensiva terroristica, cercando di screditare la controparte; ma in questo scontro il vero rischio siamo noi Consiglio, noi siamo gente seria, non siamo tra coloro che tifano per lo straniero per meschini interessi di bottega. Lei ha il dovere di unire il Parlamento e il Paese. Se intraprenderà una strada seria e responsabile, a difesa della pace e della stabilità dell'area, che è seriamente minacciata, a difesa degli interessi dell'Italia, su quella strada, signor Presidente, ci incontrerà.

presidente Conte, il Governo italiano, l'Unione europea, l'ONU, gli Stati Uniti, la Russia (mi riferisco a tutti i principali attori della comunità internazionale), ebbene tutti, seppur non con la stessa forza e convinzione, hanno chiesto al generale Haftar di fermare immediatamente la sua offensiva militare. Questi appelli sono rimasti inascoltati. Appare ormai evidente che Haftar, rinnegando gli impegni precedentemente assunti per favorire un processo politico di riconciliazione e riunificazione nazionale, punti a conquistare con la forza Tripoli, abbattendo il Governo di al-Sarraj riconosciuto dalla comunità internazionale. La Libia sta sprofondando in una guerra civile che ha già provocato centinaia di morti e migliaia di sfollati; e finora si è combattuto in aree poco popolate e con un limitato uso di aviazione e artiglieria pesante. Sappiamo tutti che, se i combattimenti non si fermeranno e coinvolgeranno aree urbane più densamente popolate e se entreranno in azione armamenti più letali, l'attuale emergenza si trasformerà in una catastrofe umanitaria di proporzioni inimmaginabili. Da un giorno all'altro ci potremmo ritrovare una nuova Siria sull'uscio di casa, con un esodo biblico di centinaia di migliaia di profughi in fuga nel Mediterraneo; e vi assicuro che, in uno scenario così, nessun porto chiuso o direttiva ministeriale potrà fermare questo flusso. Pensate poi all'altro aspetto fondamentale in questa circostanza, quello della sicurezza. I terroristi appartenenti alla variegata galassia dei gruppi radicali della regione nel caos libico avrebbero sempre più vita facile, godendo di un contesto ideale per far prosperare i vari traffici illeciti che sono linfa vitale per finanziare le loro attività. In questa prospettiva riorganizzarsi, anche al fine di lanciare attacchi verso l'Europa, sarebbe per loro una via straordinariamente semplificata. Senza contare inoltre il rischio di perdere l'accesso a risorse energetiche di importanza strategica anche per il nostro Paese. Uno scenario catastrofico, che va assolutamente scongiurato. presidente Conte, se le interlocuzioni diplomatiche e governative di cui ci ha appena riferito non riusciranno a fermare subito Haftar, sarà necessario intraprendere azioni più decise per imporre il rispetto del diritto internazionale e il ripristino della pace e della sicurezza in Libia, azioni che necessariamente dovranno coinvolgere le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'Unione africana e la Lega araba. I senatori del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto delle prerogative del Governo, auspicano che l'Italia presenti quanto prima al Consiglio di sicurezza dell'ONU una bozza di risoluzione che non solo imponga alle parti in conflitto un immediato cessate il fuoco, ma approvi anche l'invio in Libia dei caschi blu, di una missione di pace - a guida italiana e a larga partecipazione africana e araba - che vigili sul rispetto della tregua e faciliti la riconciliazione nazionale. L'alternativa a un'immediata cessazione delle ostilità in Libia, ottenuta oggi per via negoziale o domani con l'invio dei caschi blu, è una guerra dagli esiti catastrofici, non solo per il popolo libico, ma anche per il nostro Paese e per tutta l'Europa. In tal caso, per evitare un'ecatombe di civili sotto le bombe a Tripoli o sui barconi in fuga dalle coste della Tripolitania e per evitare che l'Italia si trovi ancora una volta da sola a far fronte a una situazione che sarebbe ingestibile e potenzialmente esplosiva, sarà indispensabile un corridoio umanitario, anzi, europeo, anzi, necessaria una grande operazione di soccorso umanitario che coinvolga ONU, Unione europea, Stati Uniti, Unione africana, Lega araba e Russia per attivare dalle coste libiche un ponte aereo e navale che consenta di portare in salvo i profughi libici in tutti i Paesi europei, nessuno escluso, così come in tutti i Paesi africani e arabi in grado di garantire rifugio anche solo a una piccola frazione di cittadini libici. Se la comunità internazionale non sarà in grado di impedire che la Libia risprofondi nel caos dovrà almeno farsi carico delle conseguenze umanitarie del suo fallimento. Tale fallimento non potrà essere imputabile al Governo italiano, che sta facendo ogni sforzo possibile per salvare la Libia e porre rimedio agli errori di altri Paesi e di precedenti Governi. Presidente, la ringrazio per link apre una nuova finestra"). Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:* «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi